Onorevole Presidente, La informo che in data odierna, tenuto conto del voto espresso dal Senato della Repubblica, ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni del Gabinetto da me presieduto. Il Presidente della Repubblica ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Onorevoli colleghi, è pervenuto il seguente decreto: «Il Presidente della Repubblica VISTO l'articolo 88 della Costituzione; SENTITI i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; DECRETA: Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 6 febbraio

secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari. Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo. Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta. Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa qualunque ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati. Infine, il regime di *prorogatio* del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento di atti relativi agli *interna corporis* dell'Assemblea. Passiamo ora al calendario dei lavori dell'Assemblea. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente. Il calendario dei lavori e conseguentemente l'ordine del giorno di oggi pomeriggio sono integrati con l'esame del decreto-legge sull'accorpamento delle elezioni politiche e amministrative, approvato della Camera dei deputati. Anche per questo ultimo provvedimento, che sarà esaminato come primo punto dell'ordine del giorno di oggi, si è proceduto alla ripartizione dei tempi fra i Gruppi. Trattandosi di materia elettorale, il voto finale avrà luogo con la presenza del numero legale. Rimangono inoltre in calendario gli altri due decreti-legge approvati dalla Camera dei deputati: quello in materia di missioni internazionali, che sarà esaminato subito dopo il decreto elettorale, e il decreto-legge recante proroga di termini, che sarà discusso successivamente. Alle ratifiche già indicate nel calendario precedente si aggiunge quella trasmessa dalla Camera dei deputati relativa alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Il calendario è infine integrato con la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni sollevato dal tribunale di Milano. Onorevoli colleghi, il 6 febbraio appena trascorso ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Amintore Fanfani, uno dei padri politici della nostra Repubblica. Lo ricordo oggi in quest'Aula perché l'interruzione anticipata della legislatura ci vede riuniti solo oggi per l'esame di atti urgenti e non rinviabili. La sua figura è fra quelle che certamente rimangono vive e forti anche nella nostra vita pubblica contemporanea. Il suo pensiero e il suo contributo politico sono stati per lunghi decenni continui ed intensi e hanno lasciato un segno profondo. Fanfani fu uno studioso di economia e dei rapporti di questa con l'etica e con la società. Alcune sue idee sui limiti del capitalismo contemporaneo, elaborate negli anni '30, anticiparono considerazioni e riflessioni di molti altri pensatori politici e sociali contemporanei. Fanfani partecipò attivamente all'elaborazione della nostra Costituzione e a lui si deve, dopo un lungo dibattito, la sintesi basilare dell'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Amintore Fanfani fu per molti anni presidente del Senato della Repubblica e si impegnò per l'organizzazione e la funzionalità di questa istituzione. L'archivio storico del Senato ha acquisito i diari di Fanfani e sta curandone la pubblicazione con l'intento di offrire a tutti importanti elementi di conoscenza di questa straordinaria personalità che ha dedicato l'intera vita al nostro Paese. Presso il Senato ci saranno perciò altre occasioni per ricordare il pensiero e l'opera di Fanfani e per additare ai giovani il suo esempio. Ricordarlo oggi non è solo segno di ritualità, pure dovuta, ma è il riconoscimento, credo anche da parte di molti che contrastarono democraticamente le sue idee, dell'impegno di un combattente sincero ed appassionato per la libertà, per la giustizia e per il progresso sociale.

Signor Presidente, desidero associarmi, a nome mio personale e del Gruppo che rappresento, al ricordo da lei espresso nel centesimo anniversario della nascita del presidente Amintore Fanfani. Come lei ha detto, è stato uno dei padri della democrazia repubblicana, un grande uomo politico, un capo storico di quello che è stato un grande partito della democrazia italiana come la Democrazia Cristiana, uno statista. Mi piace ricordarlo in questo senso nel momento in cui oggi sentiamo il bisogno di una politica che, affermando i suoi valori di appartenenza e magari tenacemente difendendoli, sia però capace di interpretare e di esprimere un bene comune, un senso alto di responsabilità e del dovere verso le istituzioni e verso il Paese. Fanfani è stato uno dei più importanti cultori di studi economici ed ha contribuito alla formazione di migliaia di giovani, allora universitari; ma egli è stato anche una figura simbolo di quel riformismo cattolico e di quella cultura cristiano-democratica che ha dato all'Italia molte ed importanti riforme. Fanfani aveva una visione moderna e, pochi sanno o fanno finta di non sapere, socialmente riequilibratrice nei rapporti tra economia, mercato, impresa e politica. era un credente laico e non percepì - questo io penso - fino in fondo, in un certo momento della storia italiana, la maturazione e i cambiamenti culturali e di costume intervenuti nella società italiana, sostenendo allora, il 12 maggio 1974, le tesi antidivorziste. Eppure quella legge era stata approvata con il contributo fondamentale, direi decisivo, di uomini ed esponenti della cultura cristiano-democratica del suo stesso partito.

sono sempre stati finalizzati alla crescita del nostro Paese. Mi permetto di affermare, Signor Presidente, che il patrimonio che Fanfani ha lasciato non è esclusivo, perlomeno io non lo considero tale, del partito e della cultura politica di appartenenza;

Ho avuto la ventura di conoscerlo personalmente e ricordo che nella primavera del 1975, poco più di trent'anni fa, in un convegno molto importante a Chianciano promosso da Fanfani, mi occupai del rapporto tra Provincia e comprensorio. Cominciò Cominciò lì, in qualche misura, il mio impegno diretto nella politica italiana e Fanfani mi sorprese per due motivi particolari: in primo che non molti gli riconoscevano, di essere straordinariamente umile nella formazione del programma elettorale della Democrazia Cristiana. Quelle furono elezioni regionali di particolare significato politico; parlo della metà del 1975, come tutti ricorderete. Soprattutto, vorrei che si ricordasse ancora oggi, e lo dico lieto di avere al mio fianco l'amico Baccini, che sta terminando una tesi di laurea proprio sul rapporto tra Fanfani e il partito, il significato profondo, democratico e popolare, che Fanfani seppe attribuire al rapporto tra la politica personale e il partito politico, come strumento decisivo del raccordo tra popolo ed istituzioni. Noi lo ricordiamo come il fondatore della Democrazia Cristiana come partito. Essa era nata prima, come una sorta di movimento di secondo grado rispetto ai movimenti della società.

questo è un fatto di enorme rilievo, perché proprio oggi è in discussione questo punto specifico, ossia se abbia senso o meno, e noi dell'UDC riteniamo che lo abbia, affrontare il problema della campagna elettorale imminente, nei prossimi impegni, nella convinzione che su partiti politici organizzati seriamente in termini popolari,

della formula «L'Italia è una Repubblica democratica», con cui si apre la nostra Costituzione. Fanfani è stato due volte Presidente del Senato, due volte segretario della Democrazia Cristiana e, per lunghi anni, senatore a vita, sempre dimostrando intelligenza e acutezza politica. Ha governato sei volte da Presidente del Consiglio ed è stato anche Ministro degli affari esteri, dell'interno, del lavoro, dell'agricoltura e del bilancio. Personalità di grandi aperture in politica estera, a metà degli anni Sessanta, venne chiamato a presiedere l'Assemblea delle Nazioni Unite, confermandosi uomo di pace e forte sostenitore di politiche concrete di solidarietà internazionale.

ispirato certamente alla dottrina sociale della Chiesa, ma anche alle più moderne correnti del pensiero keynesiano, per un'Italia che usciva stremata dalla follia della Seconda guerra mondiale? La dottrina economica di Fanfani, che per molti anni ha insegnato ai giovani la storia dell'economia, si è sempre mossa su linee di grande modernità. Sostenitore di una politica di piano e della grande programmazione economica, ha promosso con stile da riformatore il finanziamento di ingenti opere pubbliche, come volano dello sviluppo del Paese e strumento di giustizia sociale e di redistribuzione della ricchezza. Quella riformista è tuttora l'unanime chiave di lettura del grande piano Fanfani di edilizia popolare, che ha così fortemente connotato la rinascita economica dell'Italia. Ha sempre combattuto in prima persona la sua battaglia politica. A volte, è stato sconfitto, ma è sempre ritornato da protagonista sulla scena del suo partito, della politica italiana, del Parlamento e del Governo. Negli anni Sessanta, memore della degasperiana definizione della DC come «partito di centro che guarda a sinistra», con l'apertura ai socialisti, partecipa e promuove le nuove formule di maggioranza di centro-sinistra come strada per l'ampliamento della base democratica e la modernizzazione dell'Italia. In coscienza, possiamo dire che, proprio negli anni Sessanta, Aldo Moro e Amintore Fanfani, con l'esperienza del centro-sinistra, cui poi successivamente, con l'apporto fondamentale di Enrico Berlinguer, seguiranno gli anni della solidarietà nazionale, contribuirono con altri a porre le prime basi culturali e politiche del Partito democratico, cui tutti i senatori del mio Gruppo ed io oggi convintamente partecipiamo. Fanfani ha vissuto da protagonista le scelte strategiche che negli anni del dopoguerrra hanno cambiato il volto del nostro Paese: dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica all'istituzione della scuola media unica, con libri di testo gratuiti per i non abbienti, all'industrializzazione del Paese, all'avvio di tante grandi infrastrutture, a cominciare dall'Autostrada del Sole, ed alla definitiva identificazione nella RAI del servizio pubblico radiotelevisivo. Con Mattei e Vanoni sostenne la necessità di un forte intervento pubblico in economia ed in questa chiave si fece promotore di un forte ruolo dello Stato,

senatore Angius, fu il frutto di una sua consapevole obbedienza agli indirizzi della Chiesa. Oggi, ricordando quegli anni, dobbiamo pensare che quella battaglia e quella sconfitta gli dovettero costare molto, considerata la sua ben nota consapevolezza del valore dell'autonomia politica dei laici nella Chiesa cattolica. Fanfani ebbe un ruolo cruciale in politica estera. Forte sostenitore del valore dell'Alleanza atlantica e dei fecondi rapporti con gli Stati Uniti, ma anche realisticamente molto attento alle istanze che venivano dall'Est, a partire da una forte attenzione nei confronti dell'Unione Sovietica. Va letto in questa chiave il suo lavoro di mediazione fra Nasser e le potenze occidentali nella crisi di Suez del 1956 ed anche, durante la crisi dei la crisi dei missili a Cuba del 1962, il suo invito al presidente Kennedy di dismettere i missili installati in Puglia contro l'URSS. Voglio concludere, signor Presidente, con una osservazione di carattere

sono convinto che il Parlamento italiano di questo terzo millennio debba guardare con molta attenzione e ammirazione a quegli esempi d'impegno politico e sociale, di senso dello Stato, di apertura sociale che hanno caratterizzato così fortemente e così proficuamente la politica italiana del dopoguerra onorando il nostro Paese e, soprattutto, aiutandolo a risorgere al termine della più tremenda guerra del ventesimo secolo. Tra gli uomini politici che in quegli anni

Ci riconosciamo, signor Presidente, nelle parole che lei ha or ora pronunziato. Dalla Costituente alla ricostruzione e, successivamente, alla poderosa crescita industriale del nostro Paese, dalla fase politica del centrismo a quella dell'apertura a sinistra, Amintore Fanfani è stato tra i grandi protagonisti della lunga e feconda stagione democratica che ha segnato tutta la seconda metà del secolo scorso. Lungo questo arco di tempo egli ha dato contributi di portata storica allo sviluppo della nostra politica interna e della nostra politica estera. Bastino due soli esempi: il piano "Fanfani-casa", fondamentale e storica esperienza di programmazione economica del nostro Paese, e la sua lungimirante attività alla guida dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Fanfani è stato anche maestro indimenticabile di democrazia e di vita per generazioni intere di giovani cattolici italiani. Tratto principale della sua ricca personalità fu la coerenza, più di una volta pagata a duro prezzo, tra gli ideali professati, le parole e le opere. Auguriamoci che il suo esempio continui a dare frutti in tempi così bisognosi di rigore intellettuale e moralità politica. Per una singolare coincidenza, signor Presidente, il centenario della nascita del presidente Fanfani cade con il trentesimo anniversario della tragica perdita del presidente Moro. È una coincidenza che si carica di significati profondi per quanti hanno avuto la ventura di avere condiviso con entrambi questi due grandi *leader* parte importante, anzi decisiva, della loro esperienza politica. Sono certo, signor Presidente che, pur in questa situazione di crisi, ella vorrà prendere in considerazione la possibilità di predisporre gli atti perché il Senato della Repubblica, una volta ricostituito, possa celebrare degnamente anche Aldo Moro. Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale si associa alle nobili parole da lei espresse per ricordare Amintore Fanfani che per tanti anni ha presieduto anche questa Camera. Fanfani ebbe una visione politica che all'epoca fu rivoluzionaria, perché pose al centro dell'impegno del suo partito e dei Governi da lui presieduti i bisogni delle classi più povere del nostro Paese, dopo la distruzione morale e materiale della Seconda guerra mondiale. Fu *leader* di partito ma soprattutto un vero statista, che aprì il nostro Paese alla visione internazionale della politica, presiedendo non soltanto il Ministero degli esteri, ma anche l'Assemblea dell'ONU. Amintore Fanfani fu anche un convinto assertore della necessità che la pace sociale del nostro Paese venisse perseguita mediante un forte rapporto tra cattolici e laici. Il "Piano Fanfani" - è stato qui ricordato - per le case per tutti i cittadini rimane l'esempio di una grande intuizione politica che pose la gente più povera in condizione di apprezzare il Governo, la politica e lo Stato. Al centro dell'attenzione e del suo impegno furono i bisogni più impellenti della nostra comunità. In conclusione, posso dire che Amintore Fanfani è stato uno dei costruttori della democrazia del nostro Paese, nei difficili anni del dopoguerra.

concordare con quanto è stato detto in Aula nel ricordo di Amintore Fanfani, ma soprattutto sull'attualità politica dell'esempio del presidente Fanfani e chiarisce la differenza tra il *leader* politico e lo statista.

La DC, da movimento a partito organizzato, è stato uno dei motivi principali della presenza politica di Fanfani perché ha voluto, in alternativa all'organizzazione del Partito Comunista, realizzare la Democrazia Cristiana in movimento organizzato e in partito strutturato nel territorio, con le sezioni, con la partecipazione diretta dei cittadini, della Costituzione, che oggi noi vediamo leso, in particolare perché i partiti non sono ovviamente quelli ispirati da quell'articolo, cioè partiti democratici o che possono ospitare, in piena democrazia, tutti i cittadini per una selezione della classe dirigente. Per queste ragioni, bisogna ricordare oggi Fanfani e il partito, Fanfani e le riforme, come la riforma della casa, come le partecipazioni statali e la *golden share*, come contributo ad una politica economica del Paese, strutturata e non soltanto legata ad interessi particolari. l'interesse generale e il bene comune sono stati i fondamenti dell'azione politica di un grande uomo italiano, che oggi anche qui al Senato vogliamo ricordare non solo con affetto, ma anche con gratitudine per aver creato

Presidente, colleghe e colleghi, dell'azione politico-istituzionale del presidente Fanfani sì sono occupati tutti i colleghi che hanno parlato prima di me; non si può non condividere quanto hanno ricordato positivamente, con giudizi molto giusti, quindi non ripeterò le loro A noi de la Sinistra-l'Arcobaleno non piacciono però le icone e le immaginette e penso che non sarebbero piaciute nemmeno a Fanfani, che aveva, come noto, insieme a tante qualità politiche, anche un carattere assai aspro e, qualche volta, puntuto e polemico.

In un luogo nel quale insegnarono poi Vanoni e Saraceno, cioè un gruppo di economisti molto importanti, lui era uno dei più vivaci; aveva con gli studenti e le studentesse un rapporto di grande familiarità e simpatia, insomma, anche sotto questo profilo un professore non accademico, non borioso, con tutte le sue qualità umane, positive e negative. Questo atteggiamento portò anche nell'azione politica e politico-teorica. Con Dossetti, La Pira, Lazzati e Laura Bianchini, diede luogo alla «Comunità del Porcellino», un pensatoio tra i più singolari dell'inizio della vita democratica del nostro Paese, ed anche alla pubblicazione di un rivista, «Cronache sociali», nella quale, a dimostrazione del fatto che amava confrontarsi con chiunque, erano spesso ospitati Togliatti, La Malfa, Nenni, cioè tutto l'arco delle forze politiche italiane. Gli va riconosciuto in questo periodo una straordinaria vivacità di ingegno e soprattutto un coraggio dell'osare intellettuale, non preconfezionando gli esiti, usando l'intelligenza che aveva e la passione che lo animava per un confronto vero con le altre persone; era una caratteristica di questo gruppo, peccato si sia persa. Sempre per non far solo delle immaginette, voglio ricordare che invece, al momento del dibattito sul divorzio, a parte le sue ferme opinioni personali, ebbe delle cadute di stile che non si sarebbero aspettate

Devo dire invece a suo vantaggio, e sono certo di interpretarlo anche se non c'è più, che egli non avrebbe mai detto - lui che era rappresentante di un interclassismo attivo e non piattamente equilibrista - che Colaninno e un operaio della ThyssenKrupp sono quasi la stessa cosa.

Ero un liberale, come sono rimasto, e in quella posizione avevo anche un rapporto interpersonale, oltre che corregionale, con un uomo straordinario che ho conosciuto e apprezzato, pieno di *humour* e di determinazione.

esperienza, nella quale gli aspetti magistrali, oltre che politici e di carattere culturale, avevano una prevalenza su ogni altra motivazione che ci poteva vedere anche in contrasto. Questo volevo rappresentare, con nostalgia, ammirazione e riconoscenza ad un grande uomo della nostra Patria.

gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di Fanfani e del suo ruolo importante, prima nell'attività dell'Assemblea Costituente e poi nella costruzione della Repubblica, nell'attività parlamentare, nella sua funzione, a lungo, di Presidente del Senato. vorrei soltanto sottolineare (per questo ho chiesto la parola) una sua particolarità che allora mi colpì molto e che mi fa riflettere alla sua grande apertura sulle questioni di politica internazionale, in alcuni casi anche al suo coraggio.

ministro degli esteri, mi telefonò un giorno (ero a Botteghe Oscure, nella sede del PCI) per dirmi: devo andare a Mosca per firmare un accordo turistico fra l'Italia e l'Unione Sovietica, vuoi venire con me? Io allora ero presidente onorario di un'associazione turistica, l'Italturist, che era la più importante azienda turistica per i rapporti con l'allora Unione Sovietica: accettai di buon grado e feci questo viaggio. Fanfani per la verità mi fece partecipare solo a margine della trattativa, che non riguardava soltanto l'attività turistica tra i due Paesi, ma volle che sedessi con lui alla conferenza stampa conclusiva di quell'incontro,

mio caro amico e compagno che era uno dei dirigenti della sezione internazionale del Partito sovietico, il quale mi disse: ho visto sulla "Pravda" (in verità, sulla prima pagina) una fotografia in cui ti si vede a fianco di Amintore Fanfani;

di un esempio della sua apertura, della sua volontà di stabilire un rapporto per cercare di incrementare i rapporti con l'Est europeo in un processo di distensione e di cooperazione internazionale. Probabilmente era anche desideroso di far conoscere ai sovietici, che io conoscevo bene, che lui era amico di molti comunisti; sappiamo quanto era sottile l'ingegno di Amintore Fanfani.

senatori, mi associo volentieri anch'io a nome del Governo al ricordo di una personalità tra le più eminenti della storia della nostra Repubblica. Come è stato ricordato, Amintore Fanfani fu un autorevolissimo studioso di storia economica, deputato alla Costituente, parlamentare e *leader* della Democrazia Cristiana, nella quale iniziò la sua attività con il gruppo di «Cronache sociali»; più volte Presidente del Senato, Presidente del Consiglio, Ministro, con rilevanti responsabilità negli organismi internazionali. Si tratta sicuramente di un protagonista che ha lasciato tracce molto rilevanti nella vita politica ed istituzionale del nostro Paese, a partire dalla Carta costituzionale con il contributo alla definizione dell'articolo 1 che ella, signor Presidente, ha opportunamente sottolineato,

e partecipazione, nonché per un'attiva presenza dell'Italia sull'orizzonte internazionale in un mondo diviso e contrapposto. È ancora vivo il ricordo della sua lunga e feconda permanenza alla Presidenza del Senato al quale era molto affezionato. Molti in quest'Aula hanno potuto conoscerlo direttamente, gli sono stati amici e colleghi; molti di noi delle generazioni successive hanno avuto occasione di incontrarlo agli inizi della loro esperienza politica e ne ricordano insieme all'indiscussa autorevolezza ed anche ad una certa severità la spiccata attitudine, per molti aspetti sorprendente, al confronto con la modernità, che si lascia apprezzare ancora oggi, quando si rileggono i suoi scritti e i testi dei suoi interventi,

l'autorizzazione di chi, estraneo al Governo e al Parlamento, potrebbe essere interessato a porre il veto all'approvazione di questa normativa. Sono sicuro che il ministro Scotti si farà portavoce di questa richiesta avanzata da «la Sinistra-l'Arcobaleno».

il provvedimento in esame riguarda più specificamente la materia del procedimento elettorale e non già la materia elettorale in senso stretto perché - com'è evidente - ciò è precluso da una norma costituzionale (l'articolo 72, ultimo comma) che impedirebbe appunto che questa materia possa essere trattata attraverso la decretazione d'urgenza. Il provvedimento in esame concerne alcune questioni specifiche. alcune questioni specifiche. La prima riguarda la possibilità che nell'anno 2008 si celebrino contestualmente le elezioni politiche e le elezioni amministrative; decreto vuole garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali; intende semplificare il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero; ed infine concedere la possibilità di accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali dell'OSCE. Il presente decreto-legge, quindi, riguarda esclusivamente le elezioni del 2008, per le quali non richiede alcuna sottoscrizione per le liste che rappresentino Gruppi o partiti politici presenti almeno in una delle due Camere con due componenti di essa, o anche con due componenti del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. prevede altresì lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative, non già prevedendo la data delle elezioni amministrative, ma anticipando la finestra elettorale dal 1° aprile al 15 giugno, così consentendo di fatto la possibilità di una convocazione contestuale. I termini di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, a seguito della cessazione anticipata del mandato, è posticipato di tre giorni; il termine dell'efficacia delle dimissioni irrevocabili viene fissato al 26 febbraio 2008. l'inserimento nel turno elettorale ordinario del 2008 dei Comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, per i quali il commissariamento si concluda entro un termine antecedente a quello previsto per la votazione. Per quanto riguarda poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, si introducono alcune puntuali modifiche: si modifica la composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero, aumentando il numero dei magistrati da tre a si introduce una specifica modalità di spedizione del plico contenente il certificato elettorale; si aumenta il numero dei seggi elettorali; modificando - diminuendo, per l'esattezza il rapporto seggi-elettori; si introduce nell'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio la figura del segretario; e si elimina dal retro della scheda la dicitura «firma dello scrutatore». Le modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero vengono anch'esse modificate, consentendo in particolare la possibilità di voto al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnate in missioni internazionali; si consente altresì ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la cui permanenza all'estero sia superiore a sei mesi e che siano all'estero da almeno tre mesi; la stessa cosa viene consentita ai loro familiari e conviventi. Una norma analoga - e qui voglio precisare che i tre mesi fanno riferimento esattamente a questa categoria, non ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato - vale per i professori universitari (ordinari e associati), ricercatori e i professori aggregati che si trovano in servizio presso istituti universitari o di ricerca all'estero. La presenza degli osservatori dell'OSCE viene specificamente consentita in conformità agli impegni internazionali. Come ultima modalità afferente il procedimento, si prevede l'invio da parte del prefetto al presidente della corte d'appello della designazione dei funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti al fine di partecipare ai lavori in caso di impedimento o di assenza degli altri componenti titolari o supplenti, al fine di assicurare comunque la garanzia del buon funzionamento delle commissioni elettorali circondariali. Alla Camera sono stati approvati due soli emendamenti. Uno concerne l'esonero dalla sottoscrizione delle liste, facendo riferimento all'esigenza che possa essere sufficienti ad evitare la sottoscrizione la presentazione di almeno due parlamentari, anche se uno di essi faccia riferimento alla Camera e l'altro al Senato. Infine - altro emendamento approvato alla Camera - il termine per esercitare l'opzione del voto in Italia, nel caso di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, decorre, limitatamente alle elezioni del 2008, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la particolare congiuntura in cui si trova il Parlamento, qui ad approvare decreti-legge a Camere sciolte, consente di valutare con estremo rigore la possibilità di accedere ad ipotesi emendative. In questo senso, abbiamo allacciato nella Commissione un dialogo con il Governo, affinché molte delle questioni che sono state sottoposte all'attenzione del dibattito, e che servono semplicemente ad accentuare lo scrupolo in tutto il procedimento elettorale, possano essere valutate dal Governo non solo nella sua saggezza, ma anche nell'attività che andrà in concreto a svolgere. Mi auguro che le rassicurazioni che verranno dal Governo potranno essere di soddisfazione per i colleghi; mi riferisco in particolare al collega Micheloni che ha sollevato un paio di questioni, una delle quali dichiarata

intervengo per porre in evidenza una questione molto delicata, che non ha nulla a che fare con provvedimenti riguardanti questa o quella categoria, o questo o quel territorio. Il collega Rossi ha posto in evidenza qualche tempo fa, attraverso lo strumento eccezionale dell'incatenamento, una particolare anomalia del decreto-legge che noi dobbiamo esaminare, riguardante il diritto a partecipare alla prossima campagna elettorale. Questo decreto-legge, e mi rivolgo al collega Sinisi, tratta la materia elettorale in quanto non contiene solo norme procedurali. Vi è la materia elettorale, e la raccolta delle firme è essenziale per la partecipazione alle elezioni. Questo decreto-legge, per circostanze non facilmente comprensibili, prevede che il numero ridotto di firme necessarie per presentare le candidature sia consentito a Gruppi che abbiano due parlamentari.

Signor Presidente, non vi è nessuna ragione al mondo per la quale si debba fare un favore a chi ha due parlamentari (uno in ciascuna Camera). Infatti, o noi riteniamo che basti la presenza in Parlamento di un Gruppo politico per potersi avvalere della riduzione del numero di firme oppure stiamo violando un diritto fondamentale di eguaglianza. È bene ribadire che, per quanto riguarda l'UDC, il problema non si pone. abbiamo presenze numerose in entrambe le Camere (e quindi il problema non ci riguarda, neanche indirettamente) ma, in questo momento, non è in oggetto la convergenza o meno con le opinioni politiche del senatore Rossi (che sono lontanissime dalle nostre). Vi è convergenza, invece, sul diritto essenziale alla partecipazione alla competizione elettorale. Per questa ragione invito il Governo (che ripetutamente ha fatto capire che l'altra Camera non avrebbe fatto in tempo a convertire il decreto-legge, se modificato) a far capire che non esistono comodità di parlamentari, in tempi nei quali vi sono grandi manifestazioni popolari contro i privilegi dei parlamentari, che possano indurre il Governo a far finta di non capire

il decreto. In questo momento chiediamo, attraverso la modifica del decreto-legge venuto all'esame dell'Aula, che sia prevista espressamente la possibilità o che il decreto sia lasciato decadere allora varranno le regole in atto che sono regole di eguaglianza e, da questo punto di vista, non vi sarà alcun privilegio per nessuno) oppure che il decreto venga corretto prevedendo che basta la presenza in un solo ramo del Parlamento perché il Gruppo politico possa avvalersi dei privilegi che il decreto consente. Opinando diversamente, ed è opportuno che i colleghi se ne rendano conto, noi contravveniamo ad una specifica indicazione del Capo dello Stato che ha espressamente detto che i decreti-legge in periodo elettorale hanno senso se vi è unanime convergenza sul testo medesimo

i vari Gruppi politici dell'opposizione hanno dato il loro consenso all'abbinamento delle due tornate elettorali. Il consenso era necessario - ripeto - perché il Capo dello Stato aveva detto che senza unanimità politica ed istituzionale il decreto-legge non si sarebbe potuto adottare. Quello che ci viene dalla Camera è privo del presupposto dell'unanimità che ripetutamente il Capo dello Stato ha chiesto. Per questa ragione il mio intervento in questo momento serve ad attirare l'attenzione dei colleghi su un punto fondamentale di questo decreto-legge. Chiediamo che il Senato lo modifichi per ripristinare il principio di eguaglianza, che è fondamentale in materia elettorale, e che il Governo non si assuma la responsabilità di affermare che non vi è il tempo per convertirlo in legge perché il tempo vi è ed è abbondante; si convochi la Camera dei deputati per approvare la modifica. A quel punto vedremo quale Gruppo politico e quali parlamentari si sottrarranno all'obbligo di approvare il decreto-legge come richiesto; evitiamo di dare la sensazione, ancora una volta, che in questo Parlamento siamo soltanto attenti agli interessi delle parti politiche più forti perché in questa campagna elettorale questo è il punto che è in gioco. Non ho nulla da condividere con il collega Rossi dal punto di vista politico, ma non ho nessuna ragione al mondo per impedirgli un privilegio che viene accordato ad altri Gruppi politici

l'unanimità richiesta dal Capo dello Stato per la regolarità costituzionale - non è un fatto procedurale - e per la percorribilità politica del decreto-legge in questo senso. In questa materia abbiamo visto che la percorribilità era

Ciò che è oggi in vigore è una diversa disciplina, non vi è la discriminazione; siamo contrari ad introdurre per decreto-legge in materia elettorale, come in questo caso stiamo facendo, discriminazioni a danno di qualunque parte politica. Concludo l'intervento chiedendo al relatore Sinisi e al Governo di dare parere favorevole alla modifica di questo decreto-legge perché si raggiunga l'unanimità. Se l'unanimità non si raggiunge per la perversa volontà del Governo sarebbe molto grave che un Esecutivo dimissionario in campagna elettorale

così come al Senato chiede questo, alla Camera sarebbe presente per garantire la conversione del decreto‑legge. Evitiamo che il Governo in questo momento si assuma una responsabilità gravissima in campagna elettorale; una simile violazione da parte della maggioranza politica che approva questo decreto‑legge e da parte del Governo Non è una minaccia di alcunché; è soltanto un preannuncio di denuncia continua da parte nostra della volontà incostituzionale di questa maggioranza e di questo Governo nei confronti dei Gruppi di opposizione non graditi alla maggioranza medesima.

a determinate categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero, a cominciare dal personale diplomatico, dal personale militare in missione, nonché da insegnanti che abbiano certi requisiti e che si trovino a svolgere le loro mansioni all'estero, di un passo ulteriore rispetto a quanto avvenne due anni fa quando fu approvato un decreto di analogo contenuto in virtù del quale per la prima volta queste categorie ebbero la possibilità di esprimere il loro voto. Mentre allora, per ragioni tecniche, non si riuscì a trovare altra soluzione se non quella di farli votare come italiani residenti all'estero, partecipando perciò all'elezione di quei

per le elezioni dei deputati e senatori che si eleggono in Italia. Il secondo punto che vorrei affrontare riguarda la materia sulla quale ho presentato l'ordine del giorno G1. Noi sappiamo quello che è successo nell'elezione di due anni fa quando ci sono state, da entrambe le parti, delle contestazioni della validità dei risultati. Io vorrei attirare l'attenzione su un punto specifico della legge che deve essere rispettato per dare la massima trasparenza, affidabilità e

del Testo unico delle leggi elettorali, cioè che le schede devono essere estratte dall'urna una per volta e solo una volta che è stata assegnata una scheda può essere estratta un'altra scheda. Noi sappiamo da molte testimonianze, addirittura da fotografie che vengono pubblicate su giornali, che questo in molti casi non avviene. Si prende l'urna, la si rovescia, si fanno i cosiddetti mucchietti, uno per partito, e poi si conta. Non è la procedura prevista dalla legge e può dare luogo ad atti a quel punto sostanzialmente oltre che formalmente illeciti, che consistono, ad esempio, nel trasformare una scheda bianca in una scheda validamente votata per un partito oppure nell'annullare una scheda validamente votata per un partito aggiungendo un altro segno. Credo che la pratica del non seguire le prescrizioni dell'articolo 68 vada ricordata. Molti la mettono in atto pensando che sia la procedura corretta. Non è così: è una procedura che può dare luogo a strascichi, a dubbi, a

Questo è un punto che molto spesso non viene rispettato nonostante comporti delle precise sanzioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 104 del Testo unico, che A tal fine ho preso atto delle osservazioni fatte dal relatore e sono disposto a sopprimere la premessa del mio ordine del giorno, modificando di conseguenza la seconda parte,

il diritto costituzionale di elettorato attraverso una serie di misure che riguardano o categorie specifiche come quella degli italiani all'estero, o la categoria dei nostri militari

prevedendo sostanzialmente la possibilità, attraverso lo slittamento della finestra elettorale, di un futuro accorpamento delle elezioni politiche con le elezioni amministrative. In tal modo si realizza una misura di organizzazione che è anche ispirata ad esigenze di razionalizzazione economica e alla necessità di unificare l'utilizzazione

la questione degli emendamenti, non posso che rifarmi a quanto già detto dal relatore e ricordare le obiettive difficoltà di ulteriori percorsi emendativi. Sono state comunque già avanzate e prese le opportune iniziative, in sede di Commissione, per tener conto di molti dei valori e delle esigenze perseguite attraverso emendamenti da trasformare in appositi ordini del giorno perché l'amministrazione possa assicurare, con la propria cooperazione, le esigenze rappresentate attraverso quegli emendamenti. Per tutte emendamenti. Per tutte le altre questioni, in una materia come questa che riguarda il procedimento elettorale il Governo non può che rimettersi al Parlamento per le opportune determinazioni.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 4.2 e 4.3. Esprime, altresì, parere

da me presentati sono ispirati dal lavoro fatto dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero che in modo unanime ha condiviso una serie di raccomandazioni che abbiamo presentato al Governo il 7 febbraio.

chiede di poter modificare il tagliando che accompagna il voto per corrispondenza, partendo dalle esperienze di Paesi in cui il voto per corrispondenza funziona

che appare in prima lettura una buona decisione, perché raddoppia il numero dei seggi per lo scrutinio del voto degli italiani all'estero,

occorre individuare tra 8.000 e 10.000 scrutatori per lo stesso giorno, nel solo Comune dove si svolgono gli scrutini del voto in Italia, cosa che a noi pare assolutamente impossibile: intendiamo

per due anni noi qui siamo stati oggetto di critiche, di attacchi e di messa in discussione della validità e dell'esito del voto della circoscrizione estero. Queste cose sono inaccettabili per gli italiani all'estero, perché ci hanno offesi nelle motivazioni. Nella stessa stampa italiana sono state riprese solo queste critiche o gli pseudocomportamenti ricattatori che non hanno

che purtroppo nel mondo non è delle migliori in questi tempi. Su tutti i telegiornali e su tutti i giornali del mondo circolano infatti le immagini della Campania e di strane scene che si sono vissute in quest'Aula. Chiedo che il Governo dia risposte concrete a queste nostre richieste, in modo da poter eventualmente trasformare gli emendamenti in ordini del giorno. Non posso però accettare come sufficiente la risposta che ha dato adesso il Sottosegretario.

Il primo, fra i tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare, è quello al quale fa riferimento l'emendamento 1.1. Il problema è quello del recapito delle schede per il voto degli italiani all'estero. I brogli e le incertezze che hanno contraddistinto lo scrutinio dei voti nascevano innanzitutto dal fatto che non vi fosse una verifica puntuale della consegna

alcune di queste missive sono state recuperate da chi non era legittimato e sono state utilizzate per il voto. Il Governo si è posto in parte il problema, se è vero, come è vero, che nel modificare

al «sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata». Ci si pone quindi il problema che vi sia un'effettiva consegna nelle mani del destinatario.

in maniera abbastanza limitata. Infatti, ragionare di una consegna "con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata" significa riconoscere che il sistema in sé non è affidabile. Tra l'altro, specificare «con raccomandata, ove possibile,» significa riconoscere che la consegna dei plichi contenenti le schede per consentire agli italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto avviene quanto meno in maniera caotica. L'emendamento puntuale che ho proposto invece prevede la formulazione «consegnano a mano ovvero inviano, con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l'identificazione del ricevente». Sottosegretario, il problema è proprio questo: noi, fra la partenza del plico non abbiamo assolutamente alcuna certezza. Non abbiamo nemmeno alcuna certezza che il destinatario sia quello che effettivamente procede al voto. Capisco benissimo che c'è un problema di affidabilità dei sistemi postali internazionali, oltre ad un problema economico, di costi, però è inutile che ragioniamo di una democrazia che ha i suoi costi e poi prevediamo un sistema che non offre alcuna garanzia per il voto all'estero. Lo dico sulla base di un'esperienza che tutti i colleghi della Giunta delle elezioni

che nasce purtroppo da una verifica che gli uffici e i membri della Giunta delle elezioni hanno operato circa la farraginosità e l'incompletezza di una normativa che dovrebbe essere migliorata. Comprendo

del fatto che il legislatore ha compreso quali fossero effettivamente le lacune e non potendo intervenire immediatamente, lascia questa eredità al legislatore che sopravverrà nella successiva legislatura. PRESIDENTE. Invito il relatore

sia degli emendamenti presentati dal senatore Micheloni che degli emendamenti presentati dal senatore Manzione.

Quanto invece all'emendamento 1.200, mi rendo conto che si tratta di modifiche sostanziali della normativa, ma se si intendesse trasformarlo in un ordine del giorno con cui si invita il Governo nella legislazione successiva

alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione è un'esortazione corretta e giusta e vale in tal senso anche per il collega Manzione, che ha presentato gli

fuori del suolo nazionale avvenga con metodi e criteri completamente diversi da quelli seguiti nel 2006. Non sto qui a ricordare

senza nulla togliere a questo strumento. Sappiamo benissimo che c'è bisogno di normativa cogente. Di conseguenza, invito

del voto degli italiani all'estero garantire una maggiore correttezza alle operazioni di voto, una maggiore trasparenza e una certezza di legalità. Per questi motivi il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore. Signor Presidente, la posizione del Governo è conforme a quella già esposta dal relatore.

la mancata iscrizione all'AIRE di una serie di soggetti che si trovano all'estero per compiti istituzionali non consente loro, in via di fatto, di concorrere ad esprimere il voto alle elezioni politiche nel collegio di appartenenza. La modalità operativa qui proposta per i dipendenti di organizzazioni internazionali, mutuata da quanto previsto dall'articolo 2 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i docenti universitari, consente di far confluire presso gli uffici elettorali del Lazio

che risiedono all'estero per un lavoro svolto nell'interesse del nostro Paese non consentiamo le stesse possibilità. È un'altra delle anomalie che voglio segnalare all'Assemblea ed anche su questo aspetto vorrei verificare il parere del Governo.

dalla disciplina che invece qui si intende modificare. Per questa ragione invito il collega Manzione a ritirare l'emendamento, altrimenti sarò costretto ad esprimere un parere contrario. ma vorrei ribadire il ragionamento che ho svolto. La modifica che ho proposto tiene conto di tutti quei dipendenti di organizzazioni internazionali che, pur non avendo l'obbligo di risiedere all'estero, di fatto prestano, nell'interesse del nostro Paese, la loro attività lavorativa Si tratterebbe di un'indicazione da inserire in una norma regolamentare che potrebbe dare, perlomeno, la possibilità a questi cittadini italiani che lavorano all'estero di comprendere che c'è attenzione da parte del Governo.

che, nell'interesse del nostro Paese, svolgono all'estero la loro attività, in particolare nelle organizzazioni internazionali. Signor Presidente, vorrei solo sostenere la tesi del collega Manzione e dire al relatore che ha dato una notizia non vera all'Aula, in quanto gran parte dei funzionari italiani che lavorano nelle organizzazioni italiane all'estero sono residenti in Italia e pagano le tasse in Italia. Mi pare strano che in un'occasione di questo genere si neghi il diritto di voto a chi, oltre tutto, è residente in Italia.

Presidente, in sede di discussione generale ho indicato le ragioni per le quali questo decreto‑legge contiene una disposizione gravemente lesiva del principio di eguaglianza. Insisto perché i colleghi stiano molto attenti nella votazione di questo emendamento. In sostanza, il decreto-legge che noi esaminiamo esaminiamo prevede almeno due parlamentari per poter avere un vantaggio dalla raccolta delle firme (poi si è detto un deputato e un senatore). La Camera ha già modificato il provvedimento; il Capo dello Stato ha ripetutamente affermato che in materia elettorale i decreti-legge devono avere l'unanimità.

perché nel testo del decreto-legge sembra assolutamente certo che non sia possibile aggiungere semplicemente un deputato ad un senatore: occorre che essi siano parte dello stesso Gruppo politico. Se così non fosse, sarebbe sufficiente che ci fosse un deputato qualunque che apponga la firma insieme al collega Rossi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo la posizione del presidente D'Onofrio, il quale pone il tema della sottoscrizione delle liste da parte di un solo componente della Camera e del Senato o di altra Assemblea parlamentare. Credo che vada assolutamente compresa anche la solidarietà umana che egli di fatto sta manifestando nei confronti di un collega, il senatore Rossi, che in questo momento sta portando avanti una protesta e che credo sia in un momento

I tempi per una navetta parlamentare stringono: siamo, come dicevo, a Camere sciolte. La materia che stiamo trattando è materia elettorale: apparentemente il decreto scadrebbe il 15 aprile, in realtà tratta adempimenti che devono essere immediatamente resi operativi, pena l'illegittimità delle operazioni elettorali. Per questa ragione, signor Presidente, dobbiamo fare uno sforzo affinché il provvedimento venga licenziato così com'è. Pertanto, solo per questo, chiedo al collega D'Onofrio di ritirare il suo emendamento. a lui e a quanti manifestano nei confronti del collega Rossi la giusta solidarietà umana che non posso che augurarmi che intervenga anche una solidarietà politica

Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del relatore Sinisi e trovo davvero singolare la motivazione che è stata addotta con riferimento alla richiesta di ritiro dell'emendamento o all'eventuale parere contrario. all'eventuale parere contrario. In sostanza, si sta discutendo del fatto che se una determinata lista è sostenuta da due parlamentari non si raccolgono le firme, se invece è sostenuta da un solo parlamentare le firme si devono raccogliere.

i due parlamentari si riconoscano già formalmente, con dichiarazione di appartenenza al Gruppo Misto, alla lista per la quale la deroga dovrebbe essere operata (mi riferisco alla lista del collega Rossi).

Mi rivolgo istintivamente a quella che dovrebbe essere la mia parte naturale, anche se ha votato contro tutti gli emendamenti. Avrei gradito qualche contestazione nel merito, se ci fosse stata la possibilità, non un atteggiamento supino

Ma è stata concessa rispetto a cosa? Rispetto alle elezioni politiche (mi rivolgo al rappresentante del Governo, che forse è la persona più attenta in questo momento); rispetto ad elezioni politiche che però, in qualche modo, hanno seguito un percorso fisiologico che non è stato alterato: la questione di fiducia, la votazione della fiducia, il tentativo di conferire un incarico, lo scioglimento, la votazione. Quindi c'è stata la possibilità, da parte di tutte le componenti politiche nazionali, di prevedere quale sarebbe stato l'epilogo della situazione. Pertanto, concedere una deroga rispetto alla raccolta delle firme alla politica nazionale e ai partiti nazionali è per me una cosa un po' astrusa, perché non c'è un danno non prevedibile. Il danno non prevedibile, signor Presidente, lo si registra invece per le elezioni amministrative, laddove, per i Comuni per i quali non c'era già un turno elettorale previsto, è stata disposta l'anticipazione dell'*election* *day*, che poi è stata una conseguenza della decisione del sindaco o del presidente della Provincia di dimettersi per partecipare alle elezioni nazionali. Questo combinato disposto ha compresso, per i Comuni e le Province non a turno elettorale, la possibilità di partecipare alle elezioni amministrative. Questi soggetti,

servivano a bilanciare e a concedere quel termine. Che voglio dire? Che tutte le liste civiche che avessero pensato di poter affrontare competizioni del genere si sono trovate non di fronte ad un arco temporale prevedibile e certo o ottanta giorni), ma di fronte ad un arco temporale che è stato compresso prima dalle dimissioni del sindaco, poi dall'avvicinamento dell'*election* *day* e, infine, dal fatto che le dimissioni del sindaco sono diventate immediatamente efficaci. Allora, cosa propone Una cosa semplicissima: se c'era una deroga che andava concessa per la raccolta delle firme, questa andava concessa per le consultazioni elettorali non a turno prevedibile, nelle quali effettivamente il diritto di partecipazione è compromesso; ed è più naturale che ci siano formazioni locali che vogliono partecipare alle elezioni amministrative e non che partecipano a quelle nazionali. Nei confronti di queste l'emendamento 5.1 prevede la possibilità di eliminare la raccolta delle firme; infatti, se c'è una compressione dei termini, e quindi una riduzione di un diritto effettivo di partecipazione ad una competizione democratica, è proprio quello delle amministrazioni locali non previste per la turnazione ordinaria. Questo è il senso dell'emendamento. Aspetto anche su questo di sentire il parere del relatore Presidente, il parere del relatore è contrario. Non comprendo le ragioni per cui noi dovremmo sottrarre all'obbligo di presentazione delle firme per la sottoscrizione delle candidature tutti gli enti locali in cui vi è stato uno scioglimento anticipato e tutti gli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui termine di scadenza è prima della data delle elezioni. Trovo questa norma non comprensibile anche alla luce della conoscenza della prassi nella raccolta delle firme, che avviene solitamente nelle ultime settimane prima del voto, quindi prima della presentazione delle liste, e non già con largo anticipo. Quindi, non vi è nessun nocumento ragionevole nei confronti di questi soggetti. Per converso mi chiedo, e chiedo all'Aula, quali siano gli effetti di una norma di questo genere negli enti locali, dove chiunque può presentare una candidatura senza nessun limite e obbligo di raccogliere neanche un numero minimo di firme. Quindi, avremmo degli enti locali dove, per paradosso, potrebbero esservi tante presentazioni di candidature quanti sono i cittadini residenti in quell'ente locale. Ritengo che, sia per manifesta incongruità della proposta

del Consiglio comunale prima che le dimissioni possano sostanzialmente avere il loro effetto. Non possiamo, quindi, traslare un certo tipo di termine, posto a tutela di un certo interesse, per farne derivare conseguenze sul piano delle operazioni elettorali eventualmente iniziate a seguito dell'intrapresa

oppure noi ci dobbiamo preparare alla messa in discussione della regolarità elettorale davanti a centinaia di giudici amministrativi del nostro Paese. La questione è di estrema delicatezza e se il Senato avesse votato con un voto di astensione a favore anziché contro, com'è capitato prima, vorrei far capire che è una questione dirimente della regolarità delle elezioni. e 125 voti favorevoli; ho il timore che quelli che hanno votato contro - il collega che si è astenuto non so chi sia - non abbiamo sufficientemente valutato la posta in gioco. Non è una questione di parte politica; è una questione di principio costituzionale. La mancata unanimità rende il decreto-legge in materia elettorale particolarmente carente. Stiamo molto attenti; impegniamo il Governo a fare in modo che il decreto-legge tolga questa iniquità, altrimenti prepariamoci a decine di ricorsi elettorali. È una questione di estrema gravità.

Signor Presidente, questo decreto‑legge è stato emanato sulla base di un'intesa sull'*election* *day*. Credo che sia inevitabile esprimere un voto favorevole al decreto‑legge, anche se molte norme non ci convincono e anche se siamo convinti che su alcuni passaggi si sarebbe potuto fare di più come prospettato, per esempio, da molti emendamenti che non sono stati votati solo per ragioni di tempo e non certo per ragioni di merito. voglio approfittare di questa occasione per segnalare uno dei temi che avrebbe meritato una maggiore attenzione e sul quale si sono impegnati alcuni colleghi con

si dovrà fare perché sono convinto che se i comportamenti non saranno più che trasparenti si potranno determinare quei dubbi di legittimità e di rispetto delle regole

e a prevedere la formula della circoscrizione estero fu quella che si fondava sull'impossibilità del voto per corrispondenza nel nostro ordinamento. per ironia della sorte, le leggi ordinarie senza nessun intervento di natura costituzionale su questo punto hanno previsto il voto per corrispondenza e, quindi, hanno in pratica riconosciuto la legittimità di un sistema di voto

la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Sotto il profilo della politica estera del nostro Paese, Presidente, queste missioni confermano la vocazione dell'Italia

c'é problema, Presidente. L'articolo 11 preclude all'Italia l'uso della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e anche come mezzo di soluzione delle controversie internazionali; al tempo stesso, impegna l'Italia, nell'ambito delle istituzioni multilaterali, a dare il suo contributo per la pace e la giustizia fra le Nazioni. Questa proiezione costituzionale impegna l'Italia a favore del multilateralismo che è il primo cardine storico della politica estera italiana insieme all'europeismo, all'impegno forte per la costruzione dell'Europa come unione politica, insieme all'amicizia transatlantica e insieme alla vocazione mediterranea del nostro Paese. Ebbene, questi quattro capisaldi della nostra politica estera, una politica estera di lungo periodo che scavalca i cicli politici dell'alternanza di Governo, sono in un certo senso confermati e in un altro senso messi alla prova dalle principali missioni militari internazionali di cui parla questo decreto. considerazione le tre missioni fondamentali, quella in Libano, quella in Afghanistan e quella nei Balcani, vediamo come questi quattro capisaldi della nostra politica estera siano

meno problematica sotto il profilo costituzionale e politico, anche se non dobbiamo dimenticare che nasce per aprire una finestra temporale di opportunità per rendere possibile la soluzione della crisi israelo-libanese e di quella israelo-palestinese. Sappiamo quanto sia faticoso procedere a risultati definitivi in questo campo sappiamo come il procedere del tempo stia aumentando gli elementi di preoccupazione sia di carattere politico che di carattere militare nell'area. In Afghanistan si mantiene una situazione di alta tensione sotto il profilo politico e anche sotto il profilo della sicurezza delle nostre Forze armate, come purtroppo il caso tragico della caduta di un nostro militare, vittima due settimane fa di un attentato in un contesto nel quale un nostro reparto stava svolgendo una funzione umanitaria; naturalmente a questo nostro militare va il ricordo commosso del Senato insieme al saluto alla sua famiglia. Per altro verso, c'è la situazione dei Balcani, resa più tesa dall'auto-proclamazione unilaterale d'indipendenza da parte del Kosovo, che ha visto il riconoscimento dell'Italia in un contesto certamente problematico sul piano multilaterale, perché non condiviso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In questo caso, il nostro Paese ha dovuto scegliere tra la prospettiva della solidarietà

parte delle Nazioni Unite. La politica estera del nostro Paese resta in prospettiva una politica di amicizia nei confronti della Serbia e di offerta alla Serbia di un percorso d'integrazione europea, nella consapevolezza che una soluzione definitiva al problema dei Balcani resta necessariamente quella di una costruzione dell'Unione europea e di una inclusione dell'area complessiva dei Balcani nel processo d'integrazione europea. Al tempo stesso, da parte della nostra politica estera c'è una atteggiamento di attenzione e di amicizia nei confronti della Federazione russa: il nostro Paese non vuole in alcun modo che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo possa suonare né come atto ostile nei confronti della Serbia, né come atto ostile nei confronti della Federazione russa.

Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, il disegno di legge n. 2011, n. 2011, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, chiede al Paese un sacrificio e un impegno importante, soprattutto di carattere finanziario: 1.020 miliardi di euro per l'anno 2008. Nella discussione in Commissione difesa si è detto che avremmo dovuto discutere a lungo, capire bene che cosa promuove questo questo decreto-legge, come sono andate le nostre missioni internazionali di pace e quali sono le prospettive: insomma, cosa c'è dietro l'angolo di questo importante ed imponente sacrificio economico chiesto al Paese. Ne abbiamo discusso a lungo, signor Presidente, e ci siamo detti che la conversione in legge del decreto-legge n. 8 non è soltanto volta ad assicurare, come nelle premesse, la prosecuzione degli interventi e delle attività destinate a garantire i progressi che noi ci aspettiamo nella pacificazione e nella stabilizzazione o nel miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia. Non è solo questo, signor Presidente, onorevoli colleghi: è un grande sforzo nella partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, insomma dei nostri uomini in divisa, a missioni internazionali in cui si discute di pace e di aiuto umanitario. Il testo del provvedimento è composto di otto articoli e molti sono dedicati a questa importante missione. Se oggi il Paese ha una politica estera, lo si deve a questi uomini, che, al di là di ogni immaginabile sacrificio, pagano spesso con la vita (come nel caso del nostro maresciallo Pezzullo, l'ultima vittima immolata in Afghanistan per la costruzione della pace). pace). A questi uomini spesso si danno scarse garanzie di sopravvivenza e scarse, ma indispensabili risorse per potere far sì che la loro sicurezza e la nostra stabilità vengano garantite con il necessario intervento delle istituzioni, che prevede soprattutto l'intervento delle economie. non ci sono stati danni ai nostri due militari feriti in Afghanistan è perché avevano ricevuto da poco i nuovi blindati, quelli che in caso di esplosione di ordigni rudimentali consentono la sicurezza degli operatori. Quando parliamo di risorse così imponenti, dobbiamo spiegare al Paese che, oltre alla sicurezza, è in gioco il nostro ruolo internazionale. disegno di legge n. 2011 è indicato il nostro sforzo. Si tratta di uno sforzo imponente. In termini di contribuzione di personale alle missioni internazionali, l'Italia si colloca al nono posto per operazioni a guida delle Nazioni Unite, con 2.560 militari; al secondo per operazioni sotto la guida dell'Unione Europea, con 310 militari; al quarto posto per operazioni a guida NATO, con 5.310 militari. militari. I colleghi della cosiddetta «la Sinistra-l'Arcobaleno» ci sollecitavano a scavare nel tessuto di ciò che all'estero, grazie a queste risorse, era accaduto; ebbene, gli abbiamo fatto l'elenco di quanto questo sforzo umanitario sia stato importante per l'immagine internazionale del Paese e per la sua credibilità. All'articolo 1 abbiamo sottolineato, si prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione e il proseguimento degli importanti interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia, fuori dai teatri più visibili, dove pure la comunità internazionale ha pensato spesso di fare i complimenti all'Italia e al nostro modello militare per quella cooperazione civile e militare che sta diventando perfino un modello di studio. Al di là di ciò, vi sono situazioni meno note meno importanti dal punto di vista dell'attualità, ma non meno gravi dal punto di vista del sacrificio di vite umane e della necessità di presenziare dove è messa in discussione non solo la sicurezza degli operatori umanitari, ma la stabilità e la pace e il minimo che alle popolazioni civili di quei Paesi poveri serve per andare avanti. I nostri militari costruiscono infrastrutture e in Iraq, ad esempio, dove ancora siamo presenti, l'accento cade sui settori dello sviluppo rurale, dell'agroindustria, del microcredito, della formazione.

di conciliazione e di sostegno alle nostre Forze armate e di polizia. In Libano il nostro intervento si distingue tra il canale bilaterale, che prevede interventi nei settori delle risorse idriche, nella gestione dei rifiuti, dell'energia, e il contributo umanitario *sic et simpliciter*, importantissimo. Ricordo a me stesso e a quest'Aula che i primi aiuti umanitari arrivarono dalle navi italiane, che si affacciarono all'orizzonte del porto di Beirut quando ancora infuriavano i bombardamenti. Infine, per quanto riguarda la Somalia e il Sudan, gli obiettivi prioritari per il futuro saranno il sostegno alle iniziative di pace e l'aiuto umanitario. Tutti gli interventi sono finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale. Questo è sottolineato con forza, compreso il ripristino di servizi essenziali. In seguito alle modifiche apportate dalla Camera, all'articolo 1 è stato inserito il comma 6-*bis*, che destina la somma di 100.000 euro ad iniziative di sensibilizzazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, un grande problema che causa tante vittime, soprattutto tra i bambini. soprattutto tra i bambini. L'articolo 2 autorizza lo stanziamento di fondi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, spaziando dal rafforzamento della sicurezza in Somalia e in Sudan alle spese per il mantenimento del personale italiano presso le ambasciate in Iraq e in Afghanistan,

di cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo. I Fondi fiduciari della NATO si sono dimostrati uno strumento importantissimo, nell'ambito del partenariato per la pace, che ha coinvolto persino i Paesi dell'ex blocco orientale. Il comma 3 prevede la spesa di 14.503.000 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Iraq e in Afghanistan, oltre che - come si evince dalla relazione tecnica - in Libano, dove stiamo facendo la nostra parte, con l'apprezzamento di tutti i Governi del blocco che partecipa alla missione, ma soprattutto delle Nazioni Unite. Ebbene,

la missione in Libano, la missione in Afghanistan (che comprende sia la missione ISAF, sia la missione EUPOL per la formazione di una polizia civile afgana),

ricordiamo i Balcani. Abbiamo discusso della delicatissima vicenda del Kosovo e dell'Albania, dove passano i traffici più imponenti di stupefacenti,

Siamo in Medio Oriente, ad Hebron e a Rafa, siamo in Africa, nel Darfur, nel Ciad, nella Repubblica democratica del Congo; partecipiamo alla missione delle Nazioni Unite a Cipro siamo protagonisti di programmi di cooperazione tra le forze di polizia italiana e quelle di altri Paesi, tra cui il Kosovo, la Moldova, l'Ucraina, la Bosnia Erzegovina, i territori palestinesi e perfino Haiti. Insomma, siamo nei Paesi poveri del mondo,

Siamo impegnati a rafforzare i contingenti locali, la polizia afgana, quella libanese, gli eserciti locali, affinché un giorno si possa consegnare questi Paesi poverissimi, in cui manca il necessario, alle autorità locali. Saranno missioni lunghe ed altri sacrifici saranno richiesti al Paese. Ma al di là dell'investimento economico, che quest'Aula si appresta a licenziare, e al di là dell'importanza umanitaria di queste missioni, riconosciuta a livello internazionale, ricordo che dietro questo sforzo c'è il sacrificio di circa 10.000 nostri militari,

guardano al proprio impegno non soltanto come ad una professione, ma come ad un importante impegno umanitario e di pace, nell'interesse delle popolazioni più sfortunate del mondo. in Commissione difesa si è sperimentato, insieme con la Commissione affari esteri, un percorso di condivisione importante. Abbiamo votato quasi all'unanimità e chi non ha voluto sottoscrivere lo ha fatto non perché non lo avesse fatto precedentemente in forza di un impegno politico di sostegno al Governo Prodi, ma lo ha fatto perché probabilmente - lo dico con serenità - siamo in campagna elettorale e diversificarsi è per alcune forze che hanno sostenuto l'impegno contro questi provvedimenti un obbligo di carattere politico. Il mio è un invito pertanto a rivedere le posizioni, a pensare che dietro questo sforzo vi è un grande impegno umanitario, la necessità del Paese di rinnovare la sua credibilità internazionale, del Parlamento di fare la sua parte a favore dei tanti uomini in divisa, impegnati nelle missioni a prezzo del sacrificio della vita.

di questi anni in una discussione articolata sulla politica estera del nostro Paese. Anche questa volta, purtroppo, non abbiamo avuto occasione di svolgere una disamina approfondita rispetto alla filosofia di fondo che ispira le missioni internazionali del nostro Paese ma anche rispetto alla situazione contingente sul terreno. Vorrei ricordare che in questo decreto-legge aumenta in maniera esponenziale il numero delle operazioni nelle quali l'Italia direttamente o indirettamente partecipa. Abbiamo, anche questa volta, chiesto di poter svolgere una disamina più obiettiva e accurata, una discussione articolata, punto per punto, missione per missione, perché ognuna di queste ha una sua specificità particolare. Per ognuna di queste avremmo voluto anche noi proporre una serie di raccomandazioni e di analisi, seppur critiche, che potessero comunque contribuire ad un miglioramento della presenza, del profilo del nostro Paese a livello internazionale. Questo non è stato possibile: non è stato possibile il cosiddetto spacchettamento, ovverosia discutere in maniera articolata e concreta la questione dell'Afghanistan rispetto alle altre missioni, sulle quali in buona parte abbiamo una posizione critica, ma non necessariamente di opposizione netta. Sull'Afghanistan, invece, dobbiamo sottolineare appunto la grande difficoltà nel poter contribuire ad un salto di qualità e ad una riconfigurazione della presenza italiana e internazionale del Paese. Ma a questo verrò dopo. La questione che più ci tocca di questo decreto-legge è che per la prima volta, nell'articolato e nel titolo, si osserva una simmetria tra gli interventi di cooperazione allo sviluppo e quelli militari, comunque sia di missioni internazionali che hanno a prevalenza l'uso dello strumento militare. Questo, a mio parere, è sintomo di un preoccupante cambiamento di cultura, nel quale si pratica, e purtroppo, a nostro parere, una fusione tra la cooperazione civile e le operazione militari. Di fatto, viene consolidata dal punto di vista normativo una prassi finora seguita, in particolare in Iraq o in Afghanistan, nel caso ad esempio delle PRT, *Provincial Reconstruction Team.* Team.* Il primo punto, quindi, sul quale vorrei condividere una riflessione riguarda proprio la confusione che ci si trova a dover osservare tra attività di ricostruzione, aiuto umanitario e lotta alla povertà, da una parte, e attività di controinsurgenza o di controllo militare sul territorio.

in una regione martoriata dalla guerra e dal conflitto ed anche dall'insurgenza talebana, ci dimostra che, se non si fa chiarezza sulla distinzione dei ruoli, sulla necessità di assicurare la neutralità fondamentale fondamentale degli interventi di ricostruzione umanitaria rispetto alla presenza di contingenti militari, alla fine le due cose vengono percepite come uguali. Quindi, anche chi vuole andare a fare cooperazione allo sviluppo viene visto come parte di un'occupazione militare, a torto o a ragione, e pertanto come un avversario, non come qualcuno che cerca di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Ciò ha a che vedere con i princìpi dell'aiuto umanitario, consolidati dal diritto internazionale, di neutralità, rispetto delle parti militari presenti in un teatro di guerra o, comunque sia, di conflitto e, in linea generale, anche con una sorta di riconfigurazione del mandato istituzionale e politico delle grandi istituzioni internazionali dedicate alla sicurezza, NATO *in primis*, che vorrebbe oggi in Afghanistan, e non solo, proporsi come l'unico ed esclusivo agente globale per la sicurezza internazionale.

per la prevenzione e la gestione dei conflitti e gli elementi politici di ricostruzione, cooperazione civile e anche di sicurezza, non possono essere esauriti nella discussione che oggi dobbiamo svolgere in tempi fin troppo ristretti. In merito, credo

quale modalità unica per risolvere le tensioni, sia lo strumento migliore a disposizione della comunità internazionale. tali questioni le abbiamo già sollevate in passato e le abbiamo anche cercate di rielaborare nel corso di quest'anno e mezzo di legislatura, in particolare per quanto riguarda l'Afghanistan. La nostra posizione puramente e certamente pacifista non è abbandono della responsabilità. Abbiamo voluto cercare di praticare un percorso diverso da quello che vedeva una polarizzazione tra chi chiedeva il ritiro delle truppe *sic et simpliciter,* ispirato a princìpi anche antichi di antiimperialismo o di pacifismo formale, di maniera, e chi invece voleva e vede ancora in Afghanistan il più importante banco di prova per la sopravvivenza della NATO e dell'atlantismo e quindi oggi vuole combattere in Afghanistan una battaglia per far sopravvivere modelli antichi di prevenzione di conflitti e di sicurezza dura, che fanno leva fondamentalmente sullo strumento militare. Abbiamo voluto ascoltare anche le istanze e i bisogni del popolo afgano, che ci chiede certamente sicurezza, ma non quella assicurata oggi dalla NATO o da «*Enduring* *Freedom*»; chiede un intervento più forte e articolato per quanto riguarda la ricostruzione e il soddisfacimento dei bisogni primari; un impegno per un processo diplomatico e di pacificazione, non soltanto a livello nazionale ma anche regionale. Tutto questo oggi non c'è. Abbiamo invocato e chiesto un impegno del Governo italiano per costruire le premesse o un percorso verso una conferenza internazionale di pace che potesse sciogliere i nodi che oggi causano il conflitto ed essere anche aperta ad una trattativa con le parti insorgenti che decidono di deporre le armi e di essere parte in causa per un processo collettivo, di giustizia, verità e pacificazione a livello nazionale ed anche regionale in Afghanistan. Tutto questo oggi non c'è e ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale anche il nostro sforzo per cercare di trovare una via alternativa che possa garantire l'incolumità fisica e i diritti della popolazione afgana rischia di esaurirsi in una replica, proposta oggi a noi dalla NATO e dai principali Governi che ne fanno parte, volta ad un rafforzamento della presenza militare a discapito degli altri pilastri che servono alla pacificazione in Afghanistan ed altrove. Vorrei soltanto fare un numero: oggi di un dollaro che arriva in Afghanistan da parte della comunità internazionale solo dieci centesimi vanno direttamente agli afgani. Ciò significa che la cooperazione internazionale oggi viene vista soltanto come parte di un'operazione militare che non si interroga rispetto ai bisogni effettivi delle comunità locali afgane. Lo dice in un rapporto recente un'organizzazione internazionale rinomata, Oxfam, che invita la comunità internazionale, i Paesi membri in *Afghanistan Compact*, ad ascoltare i bisogni delle comunità locali afgane, a valorizzare le capacità indigene (ossia le capacità locali), ad evitare la commistione che oggi viene praticata nei *Provincial Reconstruction Team* tra presenza militare di controinsurgenza e aiuto umanitario, anzi, Oxfam addirittura chiede una strategia di *phase out*, di uscita progressiva dei Paesi presenti in Afghanistan dalla formula del PRT.

verso una dichiarazione unilaterale di indipendenza, avallata poi anche dal nostro Governo, rappresentasse un grave precedente e potesse (e può) essere fonte di gravi sconvolgimenti o conflitti nell'area balcanica e non solo. Crediamo che quella decisione di avallare una dichiarazione unilaterale di indipendenza (sia pure poi smorzata nei toni, perché si parla di un'indipendenza sotto il controllo internazionale, di una dichiarazione non unilaterale bensì concordata) vada al al di fuori del mandato della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza, che (vorrei ricordarlo) sanciva l'intangibilità dei confini sovrani della Serbia, e soprattutto rappresenti oggi una seria penalizzazione nei confronti di un Governo, quello serbo, che cerca faticosamente di costruirsi un percorso democratico di partecipazione e vuole creare gli anticorpi verso forme di nazionalismo retrogrado. Ma soprattutto la cosa che ci preoccupa è che oggi l'Unione Europea si presenta in Kosovo con la sua più importante missione PESD (la Eulex) con un fronte non compatto, perché molti Paesi dell'Unione Europea non concordano e non riconoscono l'indipendenza del Kosovo, Kosovo, in una situazione in cui il mandato legale internazionale è molto vago, reinterpretabile in maniera soggettiva e che quindi non trova fondamento in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Insomma, a nostro parere un precedente assolutamente preoccupante. Veniamo ora un conflitto dimenticato, ci si dice, perché l'Italia si è ritirata. Ebbene, l'Italia non si è ritirata: ha ritirato i contingenti militari, ma mantiene una *task* *force* che a Nasiriya continua ad effettuare operazioni di ricostruzione ed è presente all'interno della base americana di Tallil. Anche lì, ci dobbiamo interrogare su come intervenire, su come essere presenti, con la ricostruzione e la cooperazione, in aree di conflitto: non certo affidandosi alla protezione di compagnie di sicurezza privata, come ad esempio la Aegis, da molti vista come di fatto una compagnia che opera né più né meno come una società mercenaria. Su questo avrei voluto discutere, perché non siamo assolutamente favorevoli ad un disimpegno del nostro Paese nelle aree di conflitto, ma anzi ad un maggiore impegno con gli strumenti della diplomazia preventiva, della diplomazia popolare, della ricostruzione, del rispetto e della promozione dei diritti umani.

che ha comportato l'uso di armi sofisticatissime, che probabilmente è stata anche utilizzata come campo di sperimentazione per nuovi sistemi d'arma. Oggi le informazioni che ci arrivano da quella città fantasma ci parlano di decine e decine di bambini morti in conseguenza dell'uso di queste armi letali. chiediamo con un ordine del giorno che l'Italia si impegni presso l'Organizzazione mondiale della sanità e le Nazioni Unite perché ci sia un intervento della comunità internazionale che possa rafforzare il settore sanitario ed ospedaliero, al fine di dare agli iracheni la possibilità di curare i propri figli e di comprendere come meglio assicurare il diritto all'accesso alla salute pubblica a Falluja e in Iraq. Quindi, spero, credo, sono convinto che l'ordine del giorno che abbiamo presentato verrà accolto.

crediamo che in Darfur sia invocata soprattutto una soluzione politica che rimetta al centro le relazioni eque tra province di periferia di periferia e il Governo centrale di Khartoum perché crediamo che sia necessario riconoscere il diritto all'accesso equo a risorse scarse come l'acqua e la terra.

sconvolgimenti dal punto di vista idrogeologico e rendono sempre più difficile l'accesso alle scarse risorse. È il primo conflitto - come sostiene l'ONU - generato dal debito ecologico che il nostro ricco mondo occidentale ha nei confronti del Sud del mondo.

qualche costo inutile è ancora racchiuso in questo provvedimento. Siamo perplessi nel vedere che abbiamo dimenticato dodici carabinieri ad Hebron; non capiamo il gran senso della loro presenza. per i cinque finanzieri dislocati ancora ad Haiti. Ahimè, non dobbiamo, per la pulce, dimenticare la trave. Questo ci fa fare un passo lungo e ci fa guardare il nocciolo, il contenuto, il senso globale di questo provvedimento. Ci sembrano invece molto pochi quei 67 militari dislocati in Libia per contenere i flussi migratori, in base ad un accordo bilaterale libico‑italiano. Ci sembrano pochi perché conosciamo l'entità del fenomeno e conosciamo

più sostanzioso. Non ci può sfuggire il dato politico dietro questo aspetto. Una certa sinistra fino a ieri era probabilmente vincolata ed obbligata a votare

febbraio alcuni nostri soldati, appartenenti ad una *task force* n. 45, avrebbero anche ucciso donne e bambini. Si tratta di fonti smentite dal sistema È vero invece il contrario. Chi ha appurato, chi ha potuto confrontarsi non tanto con i nostri militari, non tanto con il sistema ISAF, ma addirittura con le istituzioni afgane, avrà potuto avere esattamente una

di altri Stati hanno una libertà maggiore: dove c'è il nemico che attacca, lì si è autorizzati a rispondere. I militari italiani, invece, devono reagire con una prudenza a volte eccessiva; ma questo ha premesso che non si siano mai verificati grossi incidenti dove civiliabbiano perso la vita*. Ergo*, la stessa popolazione ama il contingente italiano proprio per queste caratteristiche. Un altro aspetto che non posso sottacere

oppiacei - non devono verificarsi là dove i mezzi di sussistenza alternativi non sono sufficientemente presenti o là dove, probabilmente, non farebbero che esacerbare il conflitto*. Ergo*, lasciamoli produrre liberamente

nel campo delle missioni internazionali, pensando soprattutto all'interesse primario della sicurezza della nostra popolazione.

ha un carattere di arroganza e impedisce alla pubblica opinione di essere informata sull'andamento di operazioni delle quali, anche oggi, noi discutiamo il finanziamento. La legge è piena di garantire la copertura di iniziative sia nei confronti delle operazioni di cooperazione guidate dal Ministero degli affari esteri sia nei confronti di operazioni militari guidate dal Ministro della difesa.

(sperando che il prossimo Governo sia il nostro) si sia più puntuali nello svolgere questa attività di corretta informazione del Parlamento

è sollecitata soltanto nel momento in cui, purtroppo, vi è il sacrificio di un nostro uomo; inoltre, non conoscendo tutto l'aspetto positivo caratterizzante lo sforzo finanziario

dalla relazione tecnica, dove appare chiara l'esistenza di una disuguaglianza inaccettabile riferita ai compensi che lo Stato italiano dà ai suoi collaboratori impiegati in missioni di pace, a seconda che essi appartengano al Ministero degli affari esteri o della difesa. È veramente clamoroso il fatto che, a un certo punto, personale degli esteri che fa parte di certe missioni e che ha le caratteristiche di funzionario aggiunto amministrativo contabile o di assistente amministrativo o di collaboratore contabile o di collaboratore amministrativo amministrativo percepisca un'indennità che è superiore a quella di un generale di brigata. È incredibile che un contabile prenda tre volte quello che prende un capitano, volte quello che prende un sottufficiale, cinque volte quello che prende un finanziere. Ricordo che il finanziere normalmente è un diplomato che poi fa tre anni di specializzazione; ricordo che queste persone che indossano le stellette corrono rischi

Quindi, anche questo è un discorso che va corretto; è un discorso che denuncia una carenza di interessi nei confronti del proprio personale da parte del Ministero della difesa; lo dico perché mi auguro che nel prosieguo non si verifichi più per una questione di giustizia. un paio di considerazioni politiche prima di concludere. Il punto vero è che ancora una volta dal punto di vista politico nell'ambito dell'attuale maggioranza in liquidazione appare molto chiara una frattura fra la componente di sinistra, che anche qui ha appena espresso alcune idee, e e la componente di sinistra più moderata o centrale della ex Margherita. Questa frattura fa sì

La componente di sinistra che è abbastanza pesante ha cambiato un po' posizione; giustamente ha detto: «Noi non siamo più per un ritiro dall'Afghanistan;

Questo rivela ancora una volta una posizione, a mio parere, contraria per principio, una posizione classica e tipica del ruolo dell'opposizione, un'incapacità di fare proposte concrete e di assumersi la responsabilità della guida di un Paese. Ecco perché piano piano la sinistra ha trascinato la parte più responsabile e moderata verso la sconfitta e il crollo del Governo. Infine, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale ancora una volta, queste missioni si caratterizzano per un impegno vero ed autentico per la pace, assumono i connotati di una forma di carità - se volete - cristiana, di una forma di soccorso e di sostegno a popolazioni meno fortunate delle nostre e sono la dimostrazione che i nostri giovani che vestono la divisa sono capaci, come ricordava Divina, di essere grandemente apprezzati nell'ambito delle operazioni che conducono e dalle Nazioni che ne usufruiscono. Tutto ciò dimostra ancora una volta come la cultura italiana, il coraggio italiano, il senso dello Stato italiano trionfino a dispetto di tutti coloro che sono contrari, ma che non pongono e non prospettano nessuna alternativa più efficace di quella che il nostro Paese sta conducendo.

Il fatto è che queste operazioni non sono più un evento occasionale o accidentale ma sono ormai il modo naturale, direi, con cui la comunità internazionale, e quindi anche il nostro Paese, deve corrispondere alle crisi e alla proliferazione di instabilità regionale causate dall'acutizzarsi di conflitti originati da motivazioni di carattere politico, socio-economico, etnico o religioso, particolarmente dopo la fine della guerra fredda. Perché, ci chiediamo, le operazioni costano così tanto? Direi che stiamo pagando il costo di quello che mi permetterei di definire il multilateralismo inefficace che in parte c'è stato e c'è anche Costano anche perché durano tanto: in primo luogo perché spesso mancano le soluzioni politiche delle crisi che sono all'origine delle operazioni stesse; in secondo luogo perché spesso vengono condotte con scarsa capacità di pianificazione e operativa da eserciti di Paesi non sviluppati e comunque militarmente non progrediti. Entrambi i motivi rimandano alla necessità di rendere più efficace, sia politicamente che operativamente, il multilateralismo delle Nazioni Unite. Detto questo, è chiaro che è necessario spendere meglio, se le soluzioni politiche potessero essere raggiunte più facilmente in ambito ONU, così si potrebbe destinare maggiori risorse alle iniziative in si pone fin da ora un problema drammatico di efficienza della spesa, se è vero, come ricordava oggi in Commissione il senatore Martone, che su 100 dollari investiti soltanto 10 raggiungono l'obiettivo cui sono stati destinati. Dunque si impone una riflessione attenta ed un approccio nuovo. Occorre una sempre maggiore integrazione ed una non competizione tra le componenti civili e militari: le une hanno bisogno delle altre e da sola nessuna può raggiungere il suo scopo. secondo concetto che voglio sottolineare sinteticamente è che in questa nuova fase storica anche il concetto di difesa nazionale si è per così dire adeguato alla parallela evoluzione e al cambiamento della minaccia. Oggi, come sappiamo, alle minacce di tipo tradizionale cui eravamo abituati abituati si sono aggiunte, non sostituite dico io, le cosiddette minacce asimmetriche, estremistiche e terroristiche, prevalentemente non statuali che prevalgono per intensità e pericolosità su quelle tradizionali. Le minacce asimmetriche possono maturare in situazioni di instabilità e di crisi anche molto lontane da noi ma hanno una capacità di diffondere i loro effetti in un raggio d'azione geograficamente molto vasto, hanno quindi la possibilità e la facoltà di coinvolgerci direttamente. Con ogni probabilità questo tipo di minacce dominerà ancora lo scenario strategico, rallentando ed ostacolando la pacifica convivenza fra i popoli, le possibilità di sviluppo delle culture e delle economie di quasi tutti i Paesi, incluso il nostro. Questo, a mio giudizio, rende chiaro come per noi la partecipazione alle missioni internazionali e alla stabilizzazione di aree di crisi corrisponda sia ai nostri obblighi nei confronti della comunità internazionale, in conformità al dettato della Costituzione, sia ad un concetto per così dire complementare avanzato di difesa nazionale: contribuendo alla stabilizzazione dei teatri in cui siamo impegnati (dal Kosovo, al Libano, all'Afghanistan, per citare i più importanti), noi tuteliamo quei popoli e contemporaneamente difendiamo noi stessi. Non vedo quindi nessuna contraddizione tra la difesa e le operazioni che svolgiamo nelle situazioni di crisi internazionale. In terzo è proprio per affrontare con successo questi obblighi che le Forze armate si stanno progressivamente adattando alle nuove modalità d'impiego ed alle necessarie caratteristiche di interoperabilità. interoperabilità. Prima di affrontare l'esame analitico delle missioni, per il quale mi rimetterò al testo scritto, nelle quali l'Italia è presente, voglio però affrontare un punto che ha già costituito motivo di discussione nell'esame di questo decreto-legge presso la Camera e anche in quest'Aula. Tutte le missioni nelle quali siamo impegnati hanno una solida e inappuntabile base giuridica sotto il profilo della legittimità internazionale e non ci sarebbe stato motivo alcuno per il Governo, al di là della impossibilità pratica, di scorporare questa o quella il Governo, al di là della impossibilità pratica, di scorporare questa o quella missione dal pacchetto complessivo. In tutti i teatri in cui sono presenti le nostre Forze armate, lo sono su richiesta e in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

giorni fa: la morte del maresciallo Pezzullo e l'altro incidente che ha coinvolto altri nostri militari. Credo che sia giusto che, quando affrontiamo questi temi, lo facciamo sempre con il rispetto dovuto a coloro che mettono a rischio la propria vita per rispondere ad un mandato che viene loro assegnato dal Governo e dal Parlamento. Per quanto riguarda l'Afghanistan, voglio respingere di nuovo queste considerazioni sull'uso di procedure e su attività dei nostri militari non corrispondenti al mandato ricevuto, ai *caveat* nazionali e alle regole d'ingaggio loro assegnate. È in corso però una discussione all'interno dell'Alleanza Atlantica sull'efficacia della missione e sulla necessità di una revisione anche strategica che consenta di migliorare gli obiettivi finali. obiettivi finali. Alcuni Paesi dell'Alleanza, come è noto, hanno sollecitato in varie sedi un incremento dell'impegno militare da parte dei Paesi che non hanno truppe schierate nelle regioni mediorientali. Noi abbiamo detto di no a questa richiesta, insieme ad altri nostri *partner* europei, ma vorrei dire che la dialettica interna all'Alleanza, soprattutto quando è vivace, è un fatto altamente positivo, perché tende a mettere in evidenza diverse sensibilità e punti di vista, a favorire la comprensione e la sintesi politica fra Paesi alleati, che hanno un comune bagaglio di valori e di princìpi. Non è un caso che la stessa NATO stia elaborando indirizzi che valorizzino sempre più un approccio *comprehensive* al caso afgano, in cui la cooperazione effettiva ed efficace di tutte le istituzioni internazionali (ONU, Unione Europea, Banca mondiale eccetera) è vista come assolutamente indispensabile al risultato finale, che è quello della stabilizzazione e della pacificazione di quel Paese. Questo per sgombrare il campo da una serie di preconcetti che vorrebbero la NATO militarmente e muscolarmente impegnata ad espugnare l'Afghanistan; non è così, anche se bisogna ammettere che alcune cose non vanno sempre come si vorrebbe. Ci sono stati tanti problemi, sono stati commessi degli errori e, purtroppo, a farne le spese sono state molto spesso le popolazioni civili. Termino quindi l'intervento con un invito al Parlamento, in questo caso all'Aula del Senato, ad accogliere, votando positivamente, questo provvedimento. Le nostre Forze militari sono impegnate in teatri importanti e svolgono un ruolo fondamentale all'interno della comunità internazionale. È un ruolo che ci consente anche di portare avanti quelle particolari sensibilità e posizioni posizioni di natura politica che il nostro Paese ha sempre propugnato, che molte volte sono state richiamate in Parlamento, e ci consente quindi di poter dire la nostra con autorità e con autorevolezza. Noi non siamo per il disimpegno; siamo invece per un impegno coerente nello sforzo che la comunità internazionale sta compiendo. Mi auguro che tale impegno sia suffragato dal voto più ampio possibile di quest'Aula. Chiedo

ci avviamo a stanziare per le nostre missioni all'estero 1,20 miliardi. Si tratta di un impegno consistente intorno al quale c'è il consenso unanime di questo Parlamento,

Essa è all'interno della coalizione del centro-sinistra. In altri Paesi europei essa è interna allo stesso partito della sinistra: nel *Labour Party* britannico, nella SPD, nel PSOE ci sono molti deputati che la pensano esattamente come la Sinistra-l'Arcobaleno. C'è persino qualcuno tra i cristiano-democratici tedeschi che la pensa così. Ciò è del tutto normale. Il Governo non va bene poiché la situazione in Afghanistan ha preso una piega allarmante; occorre una soluzione politica, una diversa strategia della NATO; l'Italia deve chiedere tutto ciò. Tuttavia, per parlare all'interno della NATO, l'Italia deve svolgere prima di tutto il suo dovere, deve esserci, deve mantenere i suoi impegni internazionali, non deve ritirarsi. Questa è sostanzialmente la posizione del Governo,

anno, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula si è chiesto con un ordine del giorno che si affrontasse in modo innovativo la questione dell'oppio in Afghanistan. Esiste una contraddizione clamorosa ed è sotto gli occhi di tutti. L'Afghanistan in questo momento ha il massimo di controllo internazionale e, nello stesso tempo, ha raggiunto il massimo nella produzione dell'oppio: una contraddizione veramente paradossale. Si era proposto, in via sperimentale, che la comunità internazionale acquistasse a scopo farmaceutico dei quantitativi di oppio. Questa proposta non è peregrina ed ha fatto strada nell'arco di questo anno. Nel Parlamento britannico ha trovato molte voci a sostegno. Non si è riusciti a portarla avanti fino in fondo per due ragioni evidenti: perché occorre a tale scopo un consenso generalizzato e, in secondo luogo, perché si fa osservare, giustamente, che per comperare partite di oppio in un contesto di sicurezza occorre un quadro di legalità e di controllo del territorio che, purtroppo, in Afghanistan non c'è.

Questo è un obiettivo giusto ed il Governo, nei limiti del possibile, ha fatto il suo dovere per seguire l'indicazione che veniva dal Parlamento. Sull'Iraq c'è, come tutti sanno, una conferenza internazionale: il 3 novembre si è svolta ad Istanbul, la sessione successiva si svolgerà a Kuwait City, il 21 aprile. Il formato di questa conferenza internazionale è noto: vi partecipano i Paesi del G8, cioè quelli economicamente più sviluppati, i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed i Paesi confinanti. Ad Istanbul, durante la conferenza sull'Iraq, nella riunione plenaria, io stesso ho lanciato l'idea di estendere questo formato di conferenza internazionale all'Afghanistan.

non ha dato certamente risultati pratici consistenti e tuttavia ha creato un clima migliore, ha posto intorno allo stesso tavolo e, a cena, intorno alla stessa tavola imbandita, Condoleezza Rice e il ministro degli affari esteri iraniano Motaki, ha creato un *forum* in cui almeno c'è un canale di discussione. È evidente che per l'Afghanistan i Paesi confinanti hanno un ruolo decisivo nella stabilizzazione. Sappiamo che la Cina e la Russia sono insidiati dal fondamentalismo islamico, esattamente quello che si vuole sconfiggere in Afghanistan. Sappiamo che l'Iran è stato il nemico storico dei talebani, ha il dovere di proteggere una minoranza sciita contro il fondamentalismo islamico, che in questo caso è sunnita e talebano. Sappiamo che il Pakistan e l'India sono i due convitati di pietra sulla scena afgana, afgana, che si combattono per procura all'interno del territorio afgano. Quindi, una Conferenza internazionale sull'Afghanistan è assolutamente una proposta di buon senso. In quella sede, a Istanbul, ho trovato l'attenzione, l'interesse del rappresentante giapponese, di quello tedesco e di quello canadese. Non ho trovato opposizioni nette e tuttavia questa proposta si è bloccata, perché poco dopo è stata assassinata Benazir Bhutto e si è aperta una fase di instabilità drammatica per il Pakistan. Finché tale situazione non sarà stabilizzata, è difficile immaginare una conferenza internazionale, dove - come sappiamo - il Governo di Islamabad è il pilastro principale. Per quanto riguarda il Kosovo, ho sentito in questo dibattito, sia in Aula che in Commissione, e alla Camera, tante preoccupazioni fondate, certamente, e tuttavia era difficile fare diversamente, era difficile non riconoscere il Kosovo. Adesso dobbiamo guardare al futuro. guardare al futuro. Questo significa innanzitutto recuperare il tradizionale rapporto positivo con la Serbia. È interesse nazionale dell'Italia e dell'Europa che la Serbia non sia umiliata e spinta verso posizioni estremiste. In secondo luogo, dobbiamo recuperare il rapporto con la Russia. C'è a tale proposito un paradosso assolutamente anacronistico. È finita la guerra fredda, Mosca non è più la capitale del comunismo mondiale, non ci sono più motivi strutturali di contrasto e di tensione, eppure incredibilmente sta riprendendo una sorta di guerra fredda strisciante con Mosca. Ciò nasce da errori e da incomprensioni. Uno di questi errori, a mio parere, è l'insistenza degli Stati Uniti per creare uno scudo spaziale nell'Europa orientale, che viene visto dalla Russia come una minaccia nei suoi confronti. D'altronde, dobbiamo sapere che la Russia può e deve accettare intorno a sé delle repubbliche ex sovietiche trasformate in Stati indipendenti realmente autonomi, ma non può accettare degli Stati che diventino addirittura ostili, nemici nei suoi confronti. Infine, credo che si possa concludere questo dibattito manifestando un grande motivo di soddisfazione. Ci sono state critiche, ci sono state divisioni naturalmente, diverse valutazioni, ma a 180 gradi, dalla destra alla sinistra, in questo Parlamento c'è un sentimento di orgoglio, di solidarietà per il sacrificio dei nostri soldati impegnati all'estero C'è la consapevolezza

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo». non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 4.2 e 4.3. Esprime, altresì, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

è stato l'errore commesso dal Governo italiano, che si è affrettato a riconoscere l'indipendenza del Kosovo senza

La verità è che vi è stata una richiesta pressante degli Stati Uniti d'America, che da un anno hanno fatto la scelta di voler riconoscere l'indipendenza del Kosovo

all'ispirazione di Ibrahim Rugova, ma è guidato da esponenti che fino a pochissimi anni fa erano ufficialmente definiti come terroristi. Vorrei ricordare che, se in Afghanistan viene prodotto l'80 per cento dell'oppio mondiale,

decisa non si sa bene in quale contesto internazionale e in quale quadro di legalità internazionale, ci saranno militari italiani impegnati «per il ristabilimento dell'ordine». Quindi, speriamo bene che a Mitrovica e dintorni non ci ritroveremo, dopo l'ennesima missione "umanitaria", come vengono chiamate, a dover dare una mano al completamento della pulizia etnica contro i serbi. Questa è la ragione per la quale voteremo a favore di questo emendamento ed una delle ragioni che ci portano a non condividere l'impianto complessivo del disegno di legge, nel momento in cui ci è stato impedito di avere la possibilità, come sarebbe stato giusto e come è avvenuto in altre circostanze, di votare separatamente le singole missioni.

al di là della retorica della missione umanitaria, in una scelta di guerra in Afghanistan. Contrariamente a quanto si dice, e questo ordine del giorno lo dimostra, noi non siamo affatto per abbandonare l'Afghanistan a se stesso; vorremmo però un Afghanistan in cui il Governo alleato di Karzai non condannasse a morte, dopo un processo durato quattro minuti, un giornalista perché si è permesso di scaricare da un sito

Vorremmo un Afghanistan dove non si bombardasse la popolazione civile, accrescendo l'ostilità complessiva del Paese contro di noi, considerati i bianchi. Vorremmo ricordare che nessun bianco ha mai vinto in Afghanistan. vinto in Afghanistan. Vorremmo un Afghanistan nel quale non si consentisse ai signori della guerra di coltivare liberamente l'oppio soltanto perché sono alleati con l'Occidente. Vorremmo che ci fossero le Nazioni Unite in quel Paese, con un forte mandato per proteggere i civili e per realizzare la democrazia.

Signor Presidente, voterò contro questo decreto. È una posizione

bombarda in molte occasioni i villaggi e uccide donne e uomini. È una situazione di *impasse,* riconosciuta qui, riconosciuta anche per per come funziona tutto quel Paese oggi. Dunque, avremmo dovuto decidere che l'Italia non può continuare ad avere ancora più truppe dell'anno scorso, E essere impegnata per certi versi sempre di più anche nei combattimenti militari.

Era stato detto che le nostre truppe sarebbero servite per favorire il processo di pace e soprattutto per dare la possibilità ai palestinesi di vedere riconosciuti pienamente i loro diritti... *(BrusìO dai

fare? Continuo a non condividere la filosofia e l'orientamento del Governo, espresso attraverso i suoi organi (il Ministro degli esteri e il vice ministro Intini, che è qui che si riassume grosso modo in questa considerazione: solo se siamo presenti su tutti i fronti anche dal punto di vista militare possiamo contare dal punto di vista politico. Mi pare sia un'impostazione molto sbagliata, che in realtà ci subordina ad una politica imperiale dell'Occidente, che certo non può conquistare

Abbiamo chiesto di poter votare separatamente le tante missioni, perché ognuna di esse corrisponde ad un contesto giuridico e strategico diverso e quindi si presta a diverse valutazioni; tale richiesta però non ha non ha avuto esito.La richiesta di voto separato per la missione afgana è legittima perché già nel corso della XIV legislatura l'allora opposizione del centro-sinistra chiese unanimemente ed ottenne dalla maggioranza di centro-destra lo scorporo sul voto per la missione irachena. irachena. Credo che le missioni internazionali, che rappresentano l'atto più importante della nostra politica estera di sicurezza e di difesa, debbano svolgersi sempre all'interno dei princìpi fissati dall'articolo 11 della Costituzione ed essere calibrate - come ha osservato anche il Consiglio supremo di difesa lo scorso dicembre - sulle nostre risorse e su prioritari obiettivi di breve termine di mantenimento della pace nelle aree di crisi.

Esprimemmo quel voto sulla base di un impegno assunto dal ministro D'Alema circa un mutamento che si intendeva produrre per diplomatizzare la situazione afgana; l'obiettivo era una conferenza internazionale per la pacificazione

addirittura nella direzione opposta. Oggi assistiamo ad una *escalation* in tutto lo scenario afgano: nell'ultimo anno si è verificato un inasprimento del conflitto

missione in Afghanistan sia decisiva per vincere la sfida del terrorismo. È esattamente il contrario: l'occupazione militare non è la soluzione del problema afgano, ma ne costituisce una delle cause. Il terrorismo finirà soltanto quando se ne recideranno le radici socio-politiche e ciò richiederà molto tempo e non operazioni militari. Di altro c'è bisogno: la vera guerra al terrorismo che può essere vinta non si non si conduce devastando ulteriormente i villaggi semidistrutti dell'Afghanistan, ma cancellando i debiti dei Paesi poveri, aprendo i nostri ricchi mercati ai loro prodotti di base, finanziando l'istruzione per 115 milioni di bambini nel mondo attualmente privi di qualsiasi accesso alla scuola, nonché deliberando ed attuando altri provvedimenti simili.

con la necessità di affrontare i temi dell'ambiente e delle risorse in termini di redistribuzione globale. Ma il multilateralismo deve essere coerente: il primo Paese a rifiutarlo sono proprio gli Stati Uniti.

proclamata unilateralmente. Allora, nel caso del Kosovo quel che conta è lo stato di fatto, per cui la risoluzione dell'ONU che stabilisce la sovranità della Serbia diventa carta straccia, mentre per l'Afghanistan, in cui l'occupazione militare ha effetti disastrosi, conta il richiamo al multilateralismo. Come dire, signor Presidente, due pesi e due misure. A proposito del Kosovo, notiamo un effetto domino devastante. È diventato praticamente uno stato etnico; si tratta di una regione poco più grande dell'Abruzzo, con il 50 per cento di occupazione, che vive di aiuti internazionali e di malavita internazionale (il mercato del narcotraffico, come ricordava il senatore Salvi). Credo che sia stato un errore aver proceduto al riconoscimento. Avremmo dovuto rispettare la risoluzione dell'ONU, anche perché il quadro giuridico della missione PESD, al di fuori dell'ONU, è molto complicato. Siamo di fronte ad un caso di destabilizzazione, non solo

È in atto una corsa al riarmo convenzionale e nucleare. La spesa militare mondiale raggiunge i 1.200 milioni di dollari; essa produrrebbe sicuramente migliori frutti se fosse impiegata per il riequilibrio delle risorse. Nel programma elettorale del c'è scritto che si è favorevoli ad iniziative che fermino la corsa al riarmo convenzionale o nucleare. E allora perché il PD si è opposto ai nostri emendamenti, che, conformemente al programma che ci univa tutti, erano contro il rigonfiamento delle spese per gli armamenti (il sottosegretario Forcieri lo sa), che sono state del 22 per cento in questi due anni? Perché hanno fatto accordi per il cosiddetto scudo antimissile? Hanno fatto il contrario di quello che oggi sostengono. E un nostro mite emendamento, per trasferire solo 100 milioni dai 5 miliardi di spese per gli armamenti,

le condizioni di vita e il potere d'acquisto dei lavoratori, dei pensionati e dei precari, uomini e donne. Per questo siamo per la diminuzione della spesa per gli armamenti: *welfare* contro *warfare*. Per fare questo è necessario spezzare il circolo vizioso che enfatizza l'insicurezza per vendere armi e produrre guerre. Allora - concludo, signor Presidente, e la ringrazio

Stati che violano perennemente i diritti civili, non possiamo assistere inermi a Stati che compiono genocidi o che producono ordigni di distruzione di massa. Noi siamo uno di quegli Stati che, per il livello di democrazia e di sviluppo economico, non possono chiamarsi fuori da queste responsabilità internazionali. A quali condizioni? A A condizione che i nostri militari operino nella piena sicurezza (e in questo caso ci sembra una condizione soddisfatta) e a condizione che vi sia l'avallo della comunità internazionale, delle Nazioni Unite (e in questi casi si opera fianco a fianco di tutti gli Stati chiamati a rispondere in tal senso). A queste condizioni, noi non possiamo dire no a missioni di tale natura. ribadire un'ulteriore preoccupazione: sul fronte dei flussi migratori le nostre missioni sono nettamente inferiori. Il contingente italiano è nettamente inferiore alle necessità. L'Accordo libico-italiano per frenare i flussi deve essere intensificato e la presenza di poco più di 60 militari italiani significa praticamente nulla di fronte all'entità del fenomeno. Voglio ricordare a lei, signor Presidente, e al Vice ministro ancora presente, che non riuscire a gestire flussi comporta due grossi problemi all'interno del Paese. Il primo è l'incremento della criminalità,

possiamo farci carico di una miseria infinita a livello mondiale, perché non possiamo caricare sullo Stato sociale italiano queste masse di indigenti che obbligherebbero le scarse

Questo è sicuramente un *deficit* ed un fronte per il quale dobbiamo spendere di più. Ritengo, inoltre, che i nostri militari in queste condizioni debbano essere innanzitutto ringraziati per quanto stanno facendo e sostenuti con quanto questo Parlamento può fare.

Questo atteggiamento conferma la scelta fatta sin dall'estate del 2006 quando l'UDC, caratterizzandosi come l'altra opposizione, a differenza della prima opposizione

che su talune questioni, soprattutto di politica estera, e sull'impegno dell'Italia in missioni di pace non potesse esservi una valutazione politica strumentale e che, anzi, si dovesse rispettare un criterio *bipartisan*. Adesso, giunge all'approvazione di quest'Aula un testo che unifica il rifinanziamento di tutte le missioni. Per un certo verso questa impostazione impedisce un approfondimento articolato dei risultati delle singole missioni. Per l'altro verso, però, consente di disporre di un quadro d'insieme che porta, innanzitutto, ad alcune considerazioni. *In primis*, l'impegno che l'Italia sta sostenendo anche in termini finanziari, oltre che organizzativi e militari, è un impegno sempre più consistente. In secondo luogo, tutte le missioni tendono all'autoperpetuazione. Allora, sorge la necessità di stabilire un criterio e un metodo per cui, in dipendenza di dati risultati e del tempo affrontato, si possa stabilire quando vengono meno le ragioni di talune missioni.

diviene sempre più urgente ridefinire il modulo militare. Noi abbiamo un'organizzazione militare sempre più diversa e distante dalle esigenze che poi il Paese affronta di volta in volta quando si impegna in missioni di pace. Su questo punto in verità il ministro Parisi aveva promesso all'inizio della legislatura, adesso interrotta, la presentazione di una proposta e di un progetto. Io credo che questo impegno debba essere trasferito nella prossima legislatura al Governo che verrà. Mantenere questo modulo militare e poi forzarlo all'impegno delle singole missioni provoca una serie di contraddizioni che sempre più diventano insostenibili. Un'altra osservazione riguarda soprattutto le due missioni principali: l'Afghanistan ed il Libano. Credo che per queste missioni il futuro Governo della prossima legislatura debba essere pronto ad una impostazione di linea strategica che - lo dico subito - non porta a un ripensamento e, quindi, a un ritiro dell'impegno dell'impegno in Afghanistan e in Libano; la domanda però sulle prospettive e sugli sbocchi di quelle missioni diventa sempre più incalzante. A questa domanda bisogna dare una risposta e bisogna darla in sede politica con un'iniziativa politica. Sin qui l'iniziativa politica avvistata è stata quella della conferenza di pace. Credo che oggi purtroppo con molta preoccupazione si debba riconoscere che questo strumento avvistato ed indicato probabilmente non sia più facilmente praticabile perché la conferenza di pace per l'Afghanistan richiedeva un punto fermo: il Pakistan. Oggi, in quel grande teatro, rinnovando purtroppo una quasi bisecolare vicenda storica, è aperto anche il problema del Pakistan. Auguriamoci che l'esito elettorale permetta a quel Paese di avere un Governo probabilmente di grande coalizione, ma che mantenga ferma la linea dell'impegno di contrasto ai talebani perché la missione la missione nella quale siamo impegnati in Afghanistan è una missione di contrasto ai talebani. Si può anche, com'è avvenuto nel recente passato, avanzare l'ipotesi molto probabilistica o decisamente improbabile che sarebbe anche opportuno tentare un colloquio con i talebani, ma questa ipotesi probabilmente avviene più per spinte di tipo pacifista generico che non per la convinzione politica della possibilità di superare il problema dei talebani. Il problema dell'Afghanistan continua ad essere fondamentalmente quello dei talebani. Allora, credo che con molta onestà si debba dire a noi stessi che l'impegno della missione in Afghanistan non possa venire meno e che la stessa vada ripensata anche all'interno

alla strategia politica. L'altra osservazione riguarda il Libano. Il cielo ce l'ha mandata buona perché quando il Governo ha proposto di andare in Libano c'erano molte fondate ragioni per temere che l'impegno dell'Italia in quell'interstizio fosse esposto a moltissimi rischi. Sin qui è andata bene, però francamente dobbiamo constatare che i risultati, al di là degli aspetti umanitari della missione, ancora non concorrono a determinare un superamento della situazione politica e militare che ha caratterizzato il Libano. In conclusione, ribadisco il voto favorevole dell'UDC, con l'auspicio che il Governo della prossima legislatura, in una continuità di linea di politica estera, segua dei punti di riferimento, che ormai - credo - siano diventati prevalenti per tutte le forze politiche, l'ONU,

non c'é stato un atteggiamento dell'Europa molto convergente. È bene allora essere consapevoli dell'esistenza di questi problemi e lavorarci per trovare una soluzione in positivo. Presidente, con questo mio brevissimo Grazie, dei nostri militari e civili che sono impegnati nelle missioni internazionali, in zone molto difficili e anche molto rischiose. Allora, vorrei esprimere per il sacrificio dei nostri concittadini caduti in vili attentati. Si tratta di zone rischiose e di crisi che determinano, a livello internazionale, momenti di grande instabilità. Per l'Italia

abbandonato dalla comunità internazionale, anche se quest'ultima deve affrontare l'impegno afgano con maggiore determinazione e con maggiore capacità di coordinamento. anche ad altre zone che forse sono troppo dimenticate dalla comunità internazionale, penso al Corno d'Africa, alla Somalia,

debba esprimere maggiore attenzione nei confronti di tali problemi internazionali. Il voto favorevole del mio Gruppo è per la continuità

coinvolge la responsabilità dell'Italia in sede internazionale. Ricordo che in questo momento facciamo parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

facoltà. MANTICA *(AN)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento e lo facciamo avendo mutuato, rispetto all'anno scorso, un atteggiamento diverso. Voglio dire alla collega Pisa, che si stupisce di questo mutato atteggiamento, che forse le ragioni per cui noi votiamo a favore sono ingenerate dal fatto che voi avete trovato motivi per votare contro. Ciò vuol dire che il Governo si è presentato in quest'Aula con un atteggiamento ben diverso, improntato al più grande realismo ed è su questo piano che ci siamo confrontati. I tempi sono molto brevi e cercherò di essere il più sintetico possibile. Voglio dire al sottosegretario Forcieri nel votare a favore, nel ribadire che ormai questo è un modo, forse l'unico, che resta ai grandi Paesi per fare politica estera - la presenza, cioè, nelle grandi missioni internazionali ancora una volta non abbiamo colto nelle dichiarazioni del Governo e del vice ministro Intini una verità che ci manca. Noi non crediamo che esistano solo soluzioni militari e troviamo che il Governo si sia mosso molto debolmente sul piano della ricerca di soluzioni politiche che giustificassero la presenza delle truppe italiane in questi Paesi. Lo voglio dire con grande chiarezza a proposito del Kosovo, l'unico Paese sul quale mi soffermerò: quando il Governo invoca il multilateralismo, in una polemica antica con il nostro schieramento, possiamo anche accettare questa posizione, ma allora vorremmo ricordare che una politica multilaterale presuppone, nelle sedi opportune, che il Paese (in questo caso l'Italia) difenda le proprie posizioni.

tutto il possibile in sede europea perché non si arrivasse a questa drammatica conclusione. Il fatto che abbiamo accettato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo non ci può dire solo di guardare avanti, vice ministro Intini: dobbiamo anche guardare indietro, perché il Kosovo resta una mutilazione del dritto internazionale, perché non esiste copertura dell'ONU (la risoluzione n. 1244 non parla dello *status* del Kosovo) e perché l'immagine dei carri armati italiani che difendono i santuari ortodossi in Kosovo non è certamente l'emblema di un Paese pacificato che si avvia sulla strada dello sviluppo e della democrazia. A chi pensa che questo sia un errore dell'attuale Presidenza americana e di George W. Bush, voglio ricordare che a Dayton Madeleine Albright, il Segretario di Stato di Clinton, accoglieva Tachi, attuale presidente del Kosovo, allora solo comandante di una organizzazione terroristica che era l'UCK, e lo faceva sedere fra i rappresentanti serbi, creando la famosa frattura con l'allora Governo legittimo serbo di Milosevic, che non si sedette al tavolo. Voglio dire di stare attenti a immaginare che le politiche internazionali dei grandi Paesi siano legate a personaggi o a realtà politiche: sono una strategia geopolitica e ancora una volta nel dire sì al Kosovo dobbiamo riconoscere il fallimento dell'Europa nei Balcani. La gravità della situazione è tale che credo che di Kosovo continueremo ancora a parlare, non certamente in senso positivo, ma per difendere, attraverso gli italiani, una presenza minima di una minoranza serba che rischia di essere cacciata dalle sue terre. Multilateralismo fallito nel caso del Kosovo, una situazione in Libano molto discutibile (siamo andati per aprire una finestra di opportunità, ma non mi pare che ci siamo riusciti), una presenza una presenza in Afghanistan che richiede una diversa dinamica politica e forse un diverso impegno delle nostre truppe in quel Paese. Quello che daremo stasera che guarda avanti nella continuità necessaria della politica estera, ma che non può dimenticare gli errori che questo Governo ha fatto sul piano politico.

oggi si svolge in un clima ed in uno scenario politico totalmente diversi rispetto a quelli che abbiamo vissuto nelle occasioni precedenti in questa legislatura; possiamo in qualche modo verificare come il voto libero che la Sinistra-l'Arcobaleno si accinge a dare sia in qualche modo un un sigillo ad un percorso politico che finisce qua, il fallimento di un progetto politico nato nel 1996, che con la caduta del Governo Prodi vede la Sinistra-l'Arcobaleno dissociarsi totalmente dal Partito Democratico ed essere libera di portare avanti delle posizioni che noi non condividiamo ma che sono assolutamente legittime e che sono in quest'Aula

che sostenesse il Governo nella politica estera. Un Governo che non ha la maggioranza politica in Parlamento non è un Governo che ha l'autorevolezza per guidare il nostro Paese in Italia e all'estero, un'autorevolezza che è necessaria. Finisce quindi con questo voto quella che è stata un'ambiguità presente in tutta la legislatura. Il Partito Democratico, a sua volta, è libero di fare

la necessità di dover prendere un percorso alternativo a «la Sinistra-l'Arcobaleno», la necessità di correre da soli non per scelta ma per contingenza, la necessità di cercare di trovare un percorso nuovo. Si tratta tuttavia di un percorso che non può essere considerato all'altezza di una guida autorevole del nostro Paese. Non lo è perché, quando fallisce un progetto politico, chi è responsabile di questo fallimento dovrebbe avere almeno il buon senso, e forse qualche volta anche il buon gusto, di prenderne atto. Le ricette che oggi propone in termini miracolistici non possono essere considerate in alcun modo ricette degne dell'attenzione che è giusto che i nostri cittadini e gli elettori diano; non lo sono, non possono esserlo. Per quel che riguarda perché votiamo a favore? Le ragioni rimangono le stesse: siamo convinti che sia necessario rispettare tutti gli impegni presi in sede internazionale. Il nostro Paese ha un ruolo importante nel suo passato e lo avrà ancora di più nel suo futuro. Il nostro è un impegno anche nei confronti delle nostre forze militari, che con grande sacrificio, spesso con l'estremo sacrificio, portano alta la bandiera del nostro Paese. Il nostro voto, signor Presidente, sarà quindi favorevole. Con questo voto, finalmente potremo guardare al futuro in maniera diversa.

è significativo che la storia breve della XV legislatura si avvia a conclusione con la legge sulle missioni militari. Se si rivolge uno sguardo retrospettivo alla produzione legislativa che, a fatica, è stata possibile nei margini stretti della maggioranza al Senato, che si possa convenire sul fatto che le leggi del 2006 e del 2007 sul rifinanziamento delle missioni internazionali e quella dell'ottobre 2006 sulla partecipazione italiana all'UNIFIL nel Libano, insieme alla legge che oggi è in discussione, formano una coerenza di insieme che qualifica l'opera del Governo italiano sul teatro internazionale; la qualificano in termini di politica estera, come prova concreta del ruolo italiano nel multilateralismo e in termini di politica militare, che della politica estera è, in questioni di questo genere, la proiezione necessaria. Dunque, se si scorre l'elenco delle missioni in cui i militari italiani sono impegnati in tre continenti, si nota che quasi tutte sono state avviate negli ultimi dieci anni, sul finire degli anni Novanta o agli inizi del Terzo millennio. È fuori discussione che in dieci anni la funzione delle Forze armate si è ampliata ed anche trasformata, passando dalla dottrina statica della difesa alla dottrina dinamica della sicurezza. Con ciò si sono modificate anche le forme dell'impiego compiuto nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, con un intreccio stretto fra i compiti militari ed i compiti civili. Ciò si ritrova in tutte le 27 missioni, applicato ad una pluralità di obiettivi: lotta al terrorismo, contrasto all'immigrazione illegale, addestramento di polizie ed eserciti locali, controlli di confine, protezione dei profughi e, soprattutto, mantenimento e ristabilimento della pace sotto il mandato delle organizzazioni internazionali. Tuttavia, cento del personale militare e oltre l'80 per cento degli stanziamenti si concentrano nelle due aree sismiche dei Balcani e del Medio Oriente soprattutto in Afghanistan, dove è in gioco il destino della NATO, e sul Kosovo, dove è in gioco il destino dell'Unione Europea. Nelle discussioni parlamentari del 2006 e del 2007, tutta l'attenzione era concentrata sull'Afghanistan. Oggi, un'attenzione non inferiore deve essere portata sugli eterni Balcani, che come nell'Ottocento continuano a produrre più storia di quella che riescono a consumare. L'Italia dispone di qualche titolo storico in proposito, poiché l'interesse italiano verso i problemi balcanici risale quanto meno al conte di Cavour, quando era Ministro del piccolo Regno sardo. Oggi, ciò che avviene nel Kosovo appare una catena di divisioni a raggio crescente: la divisione regionale tra serbi e kosovari, la divisione balcanica tra il Kosovo e la Serbia, la divisione europea tra gli Stati che riconoscono e quelli che non riconoscono l'indipendenza, la divisione globale fra l'America e la Russia. Grave è la responsabilità della Russia, per avere ostacolato la risoluzione sullo Stato del Kosovo, predisposta dall'inviato delle Nazioni Unite Ahtisaari. Ed ora la miccia accesa sulla polveriera balcanica peggiora le relazioni tra America e Russia, già raggelate dalla controversia sul sito polacco della difesa antimissile. Nella disgregazione di ciò che resta dell'ex Jugoslavia, al fallito protettorato delle Nazioni Unite subentra adesso il protettorato europeo, senza il quale l'indipendenza del Kosovo non potrebbe reggere. La dichiarazione unilaterale di indipendenza di un Paese che non ha sufficiente capacità di *governance* effettiva, dal momento che ha una produttività minima, un'altissima disoccupazione e anche - occorre dirlo - una diffusa criminalità e illegalità,

L'Europa, che ha accresciuto il suo ruolo nella politica estera di sicurezza, ma in forza di un Trattato ancora da ratificare, è chiamata ad un impegno straordinario qual è il controllo del Kosovo e, insieme ad esso, il processo di integrazione della Serbia. La via percorribile è soltanto quella che è stata prescelta dal Governo italiano: procedere in sintonia con Germania, Francia, Regno Unito e i Paesi del Gruppo di Contatto, preparando le condizioni perché il Kosovo possa in futuro affidare appieno alle decisioni dei suoi cittadini la propria autonomia. E il banco di prova europeo è quello di ricomporre questi nazionalismi, che sono eccitati dallo stesso processo di allargamento dell'Unione. Non c'è *exit strategy*,di fronte all'impegno per la difesa della legalità e la garanzia dei diritti umani. Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto si conclude la mia partecipazione ai lavori dell'Assemblea. Se mi è permessa una parola di congedo, voglio dire soltanto che sulle questioni internazionali, come su quelle interne, ho procurato, nel Gruppo dei Democratici, di non discostarmi mai dalla tradizione liberale, cui appartengo, e dalle idee liberali, che mi appartengono. Considero un onore avere potuto, nei limiti della mia capacità, rendermi interprete di quella tradizione e di quelle idee nel Senato della Repubblica.